Leggevo anche il mio nominativo, ma non risulto né registrato né votante. Volevo confermare il voto favorevole alla relazione del relatore e anche, con l'occasione, segnalare la criticità di un sistema elettronico che, probabilmente, presenta qualche falla.

all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario»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 finestra"). La Conferenza dei Capigruppo si è riunita ieri pomeriggio tardi e ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario della settimana corrente. L'ordine del giorno della seduta odierna prevede la discussione dalla sede redigente del disegno di legge in materia di sicurezza delle professioni sanitarie e del disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione con l'Argentina nel settore della difesa. A conclusione dei due provvedimenti, la seduta sarà sospesa fino alle ore 15. Alla ripresa dei lavori, si passerà alle deliberazioni dell'Assemblea sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione. Seguirà l'esame della relazione della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sull'emergenza epidemiologica Covid-19 per la cui discussione è stata ripartita un'ora e cinquanta minuti, in base alle specifiche richieste dei Gruppi, oltre alle dichiarazioni di voto. voto. Nella seduta di domani - che, come quella di oggi, inizierà alle ore 9,30 - sarà discusso il decreto-legge sulla parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario,

Per la discussione generale del provvedimento è stata ripartita un'ora e venticinque minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi. Il *question time*, previsto per domani alle ore 15, invece, non avrà luogo. La Conferenza dei Capigruppo è convocata alle ore 15,30 di oggi per stabilire il calendario dei lavori delle prossime

politico che possa implicare anche la votazione di un atto di indirizzo per il Governo, il tema degli atti del Comitato tecnico-scientifico che hanno ispirato i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che sono stati secretati.

Bisognerebbe capire come abbia fatto il Governo, di fronte a una sentenza del TAR del Lazio che dava la possibilità ai cittadini di poter accedere a quegli atti, a fare ricorso al Consiglio di Stato bloccando tutto fino almeno al 10 settembre. Anche questo è un elemento che non riusciamo a comprendere e a tollerare, ma indipendentemente da quella questione, che avrà il suo sviluppo con la sentenza del Consiglio di Stato, vogliamo capire: il Parlamento, i senatori e i deputati hanno il diritto di consultare quegli atti o no?

che vengano consultati perché è giusto che i rappresentanti del popolo conoscano la verità su quanto accaduto.

personali. A questo punto ci chiediamo - questa è una grande occasione - dove è finita la sinistra che amava, a livello ideologico, togliere i segreti di Stato. Dov'è quella sinistra?

a gennaio dal Ministero della salute esce un piano di emergenza che prevede tre scenari, uno dei quali molto complicato per la popolazione. Proprio per questo motivo, lo scenario è talmente disastroso che quel piano viene secretato. primo episodio molto particolare. Seconda questione: viene prorogato lo stato di emergenza con l'ultimo decreto che è stato votato qui in Aula, quando di emergenze in questo momento non ce n'è assolutamente traccia, solo per poter far conservare al presidente del Consiglio Conte i suoi poteri speciali. Terza questione: la secretazione, con il ricorso al Consiglio di Stato, degli atti del Comitato tecnico-scientifico e della Protezione civile che hanno ispirato i DPCM. Cosa c'è da nascondere?

Anche quella sui Servizi segreti è infatti una questione di equilibrio dei poteri tra maggioranza e opposizione; stiamo attenti, colleghi, perché c'è oggi un Governo e c'è un'opposizione. Domani questo tema ci sarà sempre, ci sarà sempre un Governo e ci sarà sempre un'opposizione, o almeno speriamo, a meno che non si stia andando verso la direzione di una dittatura. Noi ce lo auguriamo di sicuro, è chiaro. *(Applausi)*. Anzi, illustri personaggi ed esperti hanno detto che la dittatura non arriva mai con un solo atto, ma con una serie

dittatura sanitaria o dittatura dei tecnici. Questi tecnici consigliavano il Governo, o ordinavano al Governo? Noi questo lo vogliamo sapere. *(Applausi)*. Magari ci sbagliamo, ma tutti questi atti secretati - perdonateci - legittimano il sospetto che abbiate qualcosa da nascondere. Se uno non ha nulla da nascondere, gli atti li rende assolutamente pubblici, a partire da un piano nazionale anti-pandemia di cui non conosciamo ancora i contenuti. Vogliamo vedere i contenuti. Altro che stato d'emergenza, vogliamo il piano anti-pandemia e lo vogliamo conoscere in Parlamento. *(Applausi)*. A questo punto avete una grande possibilità per dimostrarci che stiamo sbagliando e che non volete nascondere nulla: votate a favore del calendario che proponiamo noi e giovedì pomeriggio discutiamo, magari alla presenza del Presidente del Consiglio o del ministro Speranza, di tali questioni. Almeno faremo una volta per tutte chiarezza davanti agli italiani, perché vogliamo la verità.

in realtà non si raggiunge l'obiettivo; chi non ha da nascondere, chi non deve costruire accuse inesistenti, chi non si deve difendere ha bisogno di poche parole. Se devo giudicare quello che ha fatto invece poc'anzi il presidente

Non lo si fa strumentalmente, per poter fare poi questa sceneggiata anche dal punto di vista mediatico. *(Applausi)*. Tuttavia, siccome è stata chiesta una risposta ed è stato tirato in ballo il MoVimento 5 Stelle, è giusto che il presidente Romeo abbia una risposta e non ci sottraiamo rispetto a un tema obiettivamente delicato sul quale vogliamo dire anche la nostra. Se questo - ripeto - deve essere scambiato per il fatto che da un giorno all'altro non si può

Se è bastato questo al presidente Romeo per affrontare l'argomento, contento lui contenti tutti. Se invece lo si vorrà fare seriamente, noi siamo disponibili. Ci saranno altre Conferenze dei Capigruppo, ce ne sarà una oggi e poi vedremo a settembre. Lo direi molto tranquillamente e con poche parole rispetto al fiume di parole utilizzate per affrontare questo argomento.

Riteniamo che la questione posta nella Conferenza dei Capigruppo di ieri, richiamata dal presidente senatore Romeo, sia una questione molto seria e non sfugge certo a questa maggioranza l'interesse di tutto il Paese affinché ci sia la completa trasparenza su tutti quegli atti che hanno consentito al Governo di gestire la pandemia bene, come è stato riconosciuto all'Italia da tutto il mondo. *(Applausi)*. Ci saranno le occasioni opportune, a partire dai prossimi giorni, affinché ci siano tutti gli atti a disposizione del Parlamento e non saranno certo il Partito Democratico e tutta la maggioranza a negare questa trasparenza. nessuno può dare lezioni sull'esigenza di verità, perché la verità è un patrimonio in capo ad ognuno dei senatori nel momento in cui inizia il mandato di parlamentare e quindi noi, come tutti, riteniamo che la verità su quello che è accaduto, che può essere anche una verità indotta da fatti oggettivi o da interpretazioni come la politica può richiedere, debba essere un elemento oggetto del dibattito che ci sarà in questo Parlamento anche su questi temi degli atti del Comitato tecnico-scientifico. tecnico-scientifico. Dopodiché, se invece l'intento del senatore Romeo, che ha voluto provocare questo dibattito, provando ad inserire *in extremis*, alla coda di questa settimana, un tema così delicato, era provocatorio, mi lasci dire in maniera altrettanto provocatoria che probabilmente la necessità di vedere quegli atti è più di tutti del senatore Salvini, che evidentemente senza quegli atti aveva perso completamente la bussola, dicendo un giorno di aprire tutto il Paese e l'altro giorno di chiuderlo.

da parte dei cittadini ad ottenere trasparenza e il dovere della trasparenza da parte della politica, che ci ha insegnato che la trasparenza è la cifra essenziale e irrinunciabile della politica, che ha imposto la diretta *streaming* per i propri rappresentanti e adesso non proferisce una sola parola di fronte ad un atto così grave come la richiesta da parte del Governo di non far sapere ai propri cittadini e ai parlamentari eletti dalla Repubblica cosa c'è scritto di così curioso e di così pericoloso nelle carte del Comitato tecnico-scientifico. Di cose bizzarre, curiose e singolari ce ne devono essere molte, se vogliamo commentare quello che dicono certi rappresentanti del Comitato tecnico-scientifico, che dovrebbero parlare di meno e forse studiare un po' di più, perché si avventurano in considerazioni di carattere politico del tutto estranee al loro mandato; troppe ne abbiamo sentite e viste in questi mesi. La nostra richiesta ancora una volta è molto chiara, molto semplice e molto diretta. come ha detto il presidente Conte - non è un Governo che agisce con il favore delle tenebre, allora è il momento di dissipare queste tenebre e di fare luce su tutti gli aspetti di questi mesi di *lockdown* e di lotta al Covid. Aggiungo che forse ancora più grave, anche se Non si può, anche in questo caso con il favore delle tenebre, aggiungere un comma a un decreto per prorogare

quello che è avvenuto. Adesso cominciamo a capire cosa significa la richiesta di proroga dello stato di emergenza da parte del Governo: poter fare quello che vuole, a dispetto del Parlamento, perché tutto gli è consentito con la scusa dell'emergenza e della lotta al Covid. Ma noi non possiamo tollerare che questo possa ancora accadere.

credo che si stia facendo un dibattito su una cosa che non è vera. Il Governo non ha detto che non vuole desecretare gli atti, gli atti, ma ha detto che vuole mantenere la secretazione sugli atti fino alla chiusura dell'emergenza sanitaria.

avremo la possibilità di farlo quando quegli atti, chiusa l'emergenza sanitaria, saranno desecretati. Se invece vogliamo utilizzare quegli atti per la polemica politica, abbiamo bisogno che siano desecretati oggi. Ma a noi non interessa fare polemica politica, per di più in un periodo in cui il Paese è ancora in emergenza sanitaria, seppur ridimensionata e contenuta; oggi poi c'è un'emergenza in più, quella economica. Io credo che trascinare il Parlamento in una polemica giudiziaria

Non ho capito che tipo di mercanzia voleva vendere, quindi la pregherei di lasciare concludere. Prego,

Credo che possiamo benissimo pazientare per conoscere gli atti; se ci sarà eventualmente da fare polemica politica, la faremo tutti dopo che avremo conosciuto gli atti. Nessun Governo e nessuna maggioranza vogliono tenere occultato nulla; c'è semplicemente una richiesta del Governo legata all'opportunità di evitare di desecretare gli atti fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria. Non mi sembra uno scandalo;

Devo dire che l'intervento del presidente Faraone mi ha confermato l'opportunità che il Governo riferisca e faccia chiarezza sulla questione. che gli italiani, che hanno affrontato con grandissimo senso di responsabilità e disciplina il difficilissimo e più intenso periodo della chiusura, della quarantena,

tutte queste restrizioni, con le multe, con le grossissime difficoltà economiche e con il prolungamento dello stato di emergenza fino a ottobre. Proprio perché le cose sono collegate,

parlamentari, rappresentanti del popolo, di conoscere le ragioni per le quali siamo ancora in uno stato di emergenza *(Applausi)*, uno stato di emergenza in base al quale si governa e si limitano le libertà costituzionali con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, strumento che neppure viene menzionato nella Costituzione.

A questo si aggiungono il disegno di legge, a prima firma del senatore Caliendo, sugli incarichi politici di magistrati (Atto Senato 255) e il disegno di legge per l'istituzione della «Giornata delle vittime di errori giudiziari» (Atto Senato 1686). Direi che sono temi che hanno la loro rilevanza, che coinvolgono centinaia di migliaia e indirettamente milioni di cittadini e credo che meritino l'attenzione del Parlamento in questo momento.

Il punto è il seguente. La strumentalità dipende dal fatto che ci sarebbe dovuto essere l'accordo sul calendario; è stato emesso da un giorno all'altro. che la Lega sta fuggendo dalla questione dell'autorizzazione a procedere sul caso Siri, la cui calendarizzazione

una dalla Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia; un'altra solo da Forza Italia - sulle quali si è già sviluppato un dibattito.

richiamo al Regolamento. Nello specifico, l'articolo 55 recita: «Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, possono essere avanzate proposte di modifica da parte di un senatore per Gruppo. Sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno». È evidente che ciascun senatore può presentare una proposta, come hanno fatto i senatori Romeo e Malan;

di più, non essendo dichiarazioni di voto, ma interventi sulle proposte, tantomeno è consentito un intervento in dissenso.

direi tutt'altro che trasparente nei confronti del Parlamento, è diventata un problema chiaro a tutti. È diventata un problema per quanto riguarda gli atti e, ove il Parlamento oggi prendesse una decisione diversa rispetto a quella richiesta dai Gruppi Forza Italia e Lega, noi investiremo della questione il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che, per delega del Parlamento, in questa materia ha il compito di intervenire. Mi auguro, però, che lo faccia il Parlamento.

con una votazione su una risoluzione della maggioranza. Ebbene, in quella risoluzione non c'è l'argomento poi trattato nella notte nel decreto emesso dal Governo.

Quindi il Parlamento non viene informato in via preventiva; il Parlamento non dà indicazioni di tal guisa al Governo ma il Governo, nella notte, scrive un decreto che contiene, all'articolo 1, diversi commi che modificano le procedure di nomina dei servizi segreti, tra l'altro a mio avviso - violando alcuni dettati costituzionali, e nel comunicato che illustra il provvedimento non dice nulla proprio su questo. questo. Ritroviamo così pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, all'insaputa del Parlamento, all'insaputa degli organi di informazione e dell'opinione pubblica, una norma che modifica le procedure di nomina

n. 124 del 2007, approvata da maggioranza e opposizione. Dico questo, però, perché è chiaro a tutti che c'è un problema di trasparenza e di leale collaborazione degli organi istituzionali che interferisce anche nella votazione che stiamo per fare. Mi auguro che il Parlamento - e soprattutto chi ha parlato di *streaming*, di trasparenza e quant'altro ancora - decida per la trasparenza in quest'atto.

Prego di nascondere lo striscione, che dice cosa nascondete.

in terza lettura un disegno di legge d'iniziativa governativa, che - come il Presidente ha citato poc'anzi - reca disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nell'esercizio delle loro funzioni.

apportate modifiche a mio avviso migliorative, che hanno rafforzato e implementato alcuni aspetti di rilievo, che vado ad enumerare. L'articolo 1 esplicita i richiami normativi per le nozioni delle professioni sanitarie e socio-sanitarie: come vi dicevo, è stato migliorato, perché è stata ampliata la categoria delle professioni, richiamando gli specifici articoli 4 e da 6 a 9 della legge n. 3 del 2018. L'articolo 2 prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui vi parlerò molto più approfonditamente in seguito. L'articolo 3 prevede la promozione di iniziative d'informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente le professioni sanitarie e socio-sanitarie. L'articolo 4 stabilisce pene aggravate per i casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a soggetti esercenti una delle professioni summenzionate o a soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività.

summenzionati, a causa o nell'esercizio della relativa professione o attività. L'articolo 6 esclude, nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti summenzionati nell'esercizio delle loro funzioni, i reati di percosse e lesione personale dall'ambito delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa. L'articolo 7 prevede l'adozione di misure di prevenzione - intese a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia - da parte delle strutture in cui opera il personale sanitario e sociosanitario. L'articolo 8 prevede l'istituzione della "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari". L'articolo 9 una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi di condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria o che svolga attività ausiliarie delle medesime. L'articolo 10 reca le clausole di invarianza finanziaria. colleghi, entro maggiormente all'interno di quest'articolato importante, il cui *iter* oggi porteremo a termine, facendolo diventare una legge. L'articolo 1, che - come vi dicevo - è stato inserito alla Camera, esplicita in maniera molto più appropriata l'individuazione nell'ambito delle professioni sanitarie e socio-sanitarie. trovano applicazione le norme generali in materia, in base alle quali e al relativo stato di attuazione, le professioni sanitarie sono al momento quelle riservate agli iscritti agli albi professionali dei seguenti ordini: dei medici-chirurghi degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e chimici; delle professioni infermieristiche; di quelle di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; e degli psicologi. Le professioni socio-sanitarie comprendono, in base allo stato di attuazione delle

L'articolo 2 del disegno di legge demanda a un decreto ministeriale l'istituzione, presso il Ministero della salute, del suddetto Osservatorio nazionale e la definizione della durata e della composizione dello stesso.

una relazione affinché si sappia che cosa è stato rilevato. Si prevede che ciò spetti al Ministero della salute, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, ovviamente d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni

Riguardo alla composizione dell'organismo, essa è stata migliorata e implementata. Ricordo di aver presentato emendamenti che sono stati bocciati dalla precedente

Altri rappresentanti degli ordini professionali interessati devono far parte dell'Osservatorio, oltre alle organizzazioni di settore e alle associazioni di pazienti: altro aspetto essenziale, in quanto il punto di vista dei pazienti è fondamentale.

nell'esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno ed alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro

3) che l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmetta tramite l'Agenas al nuovo Osservatorio i dati in materia acquisiti dai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente

promuovono, ovviamente, studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti.

per l'Osservatorio, ma soprattutto per la sensibilizzazione. Quindi, esprimo ovviamente tutta la mia soddisfazione per essere riusciti a portarlo a compimento in terza lettura. Devo ringraziare, in questo caso, tutti i colleghi della Commissione per essere addivenuti

che i lavori delle Commissioni di riferimento si sono svolti con la massima correttezza dei rapporti tra i Gruppi parlamentari, al fine di garantire la necessaria dialettica parlamentare e il dovuto confronto istituzionale tra Parlamento e Governo. Questo ci consente oggi di procedere all'esame conclusivo del disegno di legge in esame. Ringrazio, pertanto, a nome del Governo, i Presidenti delle Commissioni di merito; i relatori che, sia alla Camera che al Senato, si sono adoperati con il massimo livello di professionalità e competenza e tutti i componenti delle Commissioni di merito. Un apprezzamento particolare va, chiaramente, anche al lavoro degli Uffici delle Commissioni. Il disegno di legge, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, oggi qui in esame per l'approvazione finale, è stato fortemente voluto dal precedente Ministro della salute, Giulia Grillo, ed è frutto della volontà governativa di individuare misure di prevenzione e contrasto nei confronti di atti di violenza posti in essere a danno di tutti gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. concreto, predisposto dal Governo, che offre strumenti preventivi e dissuasivi e si pone l'obiettivo di incrementare la sicurezza di professionisti che quotidianamente mettono a repentaglio la propria incolumità psicofisica nello svolgimento delle loro attività. Com'è noto, si tratta di un fenomeno in crescita, aggravato ulteriormente dal fatto che, negli ultimi anni, si è assistito ad atti di particolare gravità. Non è possibile

di una sala operatoria, così come nei pronto soccorso. Le aggressioni si verificano prevalentemente nelle ore notturne. Le donne sono più colpite rispetto agli uomini e i casi sono sicuramente sottostimati. Sebbene i dati mostrino circa cinque violenze al giorno, verosimilmente tali numeri sono almeno tre volte superiori e si stima che, nell'arco della vita professionale - ad esempio - degli infermieri, circa 230.000 infermieri su 260.000 abbiano ricevuto una qualche forma di aggressione, che va da quella fisica a quella verbale. Spesso le aggressioni sono fatte da

è rallentato durante il periodo del Covid ed è ripreso subito dopo la fine dell'emergenza e la fase acuta. Non elenco i dettagli dei provvedimenti, avendo la relatrice Boldrini offerto il suo contributo, ma ci tengo a ringraziarvi per aver compreso in tutti i passaggi di questo atto in modo profondo e sincero il valore, la dedizione e il sacrificio di tutti gli operatori sanitari (medici e infermieri), che quotidianamente ci assicurano salute, ci salvano la vita e ci aiutano nel momento del bisogno. Secondo me, questo è un atto

l'aderenza ad esso da parte di coloro che vi lavorano. Cominciamo a rispettare chi ci aiuta. Lavoriamo tutti insieme per costruire una cultura di rispetto reciproco, partendo dalle Aule del Parlamento. Personale sanitario e pazienti sono entrambi dalla stessa parte; non ci dimentichiamo questo: personale sanitario e pazienti sono dalla stessa parte. Ringrazio per il vostro lavoro e mi auguro un'approvazione dell'atto all'unanimità.

signor Sottosegretario, il provvedimento che ci accingiamo a votare conclude il suo *iter* dopo quasi un anno di lavoro da parte delle Commissioni di Camera e Senato. C'è stato un dibattito molto importante che ha avuto il merito di consolidare l'impianto della legge per essere davvero uno strumento a tutela degli operatori sanitari. Le aggressioni e le violenze contro il personale sanitario sono la spia delle situazioni sociali estreme nelle quali i medici, gli infermieri, gli OSS e tutti gli operatori della sanità si trovano spesso ad operare. Non è solo questo, perché molte aggressioni nascono in un contesto di malfunzionamento del sistema sanitario. Potremmo quindi dire che il Covid ci ha solamente dato un motivo in più per consolidare l'impegno a favore dell'assistenza socio-sanitaria; strutture non fatiscenti sono strutture che proteggono il personale, ma sono anche luoghi funzionanti dove la sanità può esprimere tutta la sua efficienza, rimuovendo quindi una delle cause delle aggressioni. Un altro punto altrettanto importante è quello del presidio da parte delle Forze dell'ordine, soprattutto nelle ore notturne, nelle piccole strutture che magari agiscono in contesti periferici. Questo a tutela anche degli altri pazienti e di chi arriva in pronto soccorso, per fare in modo che non si trovino in situazioni che possano portare ulteriore danno alla loro condizione di salute. Il Gruppo per le Autonomie esprimerà quindi - come ha fatto anche in prima lettura - un voto convintamente favorevole al disegno di legge. Lo facciamo con la convinzione che questo sia un tassello di quel profondo processo di ripensamento e di rilancio del ruolo del servizio sanitario nel nostro Paese, un impegno che questo Governo ha già intrapreso nelle settimane del Covid con gli innesti di nuovo personale sanitario e le tante risorse che sono state dedicate per rafforzare le strutture chiamate a curare il virus. È un impegno - come abbiamo detto anche in altre circostanze - che dovrà continuare con grande intensità nelle settimane e nei mesi a venire, perché se c'è una cosa che ci ha insegnato la pandemia è che l'accesso universale alle cure attraverso una sanità all'altezza è un pilastro di un Paese che vuole ritenersi tra quelli più avanzati al mondo e ci ha insegnato anche il valore della nostra classe medica, degli infermieri,

un episodio gravissimo accaduto all'ospedale di Latina, sabato o domenica della settimana scorsa.

c'è anche, evidentemente, invarianza di fatti concreti e di novità rilevanti. Al di là di questo, abbiamo votato il testo, come avete visto, colleghi, semplicemente perché il più contiene il meno nella speranza che prima o poi si possa provvedere a normative certamente più stringenti e più cogenti, il Gruppo Fratelli d'Italia ha provveduto a votare un testo che contiene due due o tre cose che comunque vanno fatte e andranno fatte, non si capisce bene con quale denaro e con quali risorse, ma vedremo e giudicheremo nei fatti.

istituisce osservatori, giornate della memoria, *task force*, tutti succedanei della politica, tutte imitazioni vorrei dire cinesi - della necessità della politica di assumere decisioni importanti e quindi vie di fuga

la giornata in cui si celebra la necessità di proteggere le professioni socio-sanitarie: buoni intendimenti, ma che poco aggiungono al problema che, ripeto, è serio, reale e cogente. Ci sono alcuni passaggi positivi, come l'adeguamento delle strutture, pensare, ad esempio, alle strutture in cui solitamente sono ospitati i Sert, oppure a quelle in cui operano la generalità dei responsabili dei servizi sociali comunali.

c'è anche qualcosa che potrà un giorno rivelarsi probabilmente utile. Il problema è di carattere generale e si inquadra in un momento di

un momento in cui, evidentemente, il mondo delle professioni non riscuote la necessaria considerazione da parte dei Governi e del Governo attuale *in primis.* Rispetto a questo tema noi avevamo chiesto, come Fratelli d'Italia, sia al Senato in sede di incardinamento, sia alla Camera in sede di seconda lettura, la previsione della qualifica di pubblico ufficiale dell'esercente la professione socio-sanitaria, nel momento in cui agisce nell'orario di lavoro. È evidente la

funzione pubblica per eccellenza, cioè la tutela della salute come bene primario per la vita umana: per quale motivo non dovrebbe essere qualificato come pubblico ufficiale, con tutto quello che ne consegue in termini di repressione e di e di sanzione degli atteggiamenti di aggressività? Questa proposta non è passata, ma noi riteniamo che debba essere riconsiderata nel momento in cui finalmente si potrà affrontare

perché, signor Presidente, proprio in questi giorni abbiamo visto l'esplicarsi e il palesarsi di provvedimenti giudiziari, che avranno il loro corso e il loro esito. Io non giudico i fatti; saranno e sono sicuramente fatti penalmente rilevanti

percorsi formativi. In questa sede, noi auspichiamo e speriamo che venga prevista la possibilità che chi opera nell'esercizio di queste funzioni possa essere riconosciuto quale pubblico ufficiale, con tutto quello che ne consegue. Signor Presidente, come dicevo, io esaurisco il mio intervento e faccio recuperare un po' del tempo che aveva rubato la collega Boldrini, la quale evidentemente, dovendo illustrare il provvedimento, di maggior tempo aveva bisogno. Come si Come si è visto, noi abbiamo votato tutti gli articoli, pur avendo ampi margini di dubbio rispetto a questo testo, perché andava comunque dato un segnale a un mondo a un pezzo d'Italia che, specialmente negli ultimi tempi e nella vigenza dell'emergenza Covid-19, ha dato ottima ha dato ottima prova di sé e ha mostrato la capacità del mondo delle professioni sanitarie di affrontare le emergenze anche nel momento in cui il quadro normativo a disposizione magari non era dei dei più rassicuranti e neanche dei più protettivi, senza voler parlare dei dispositivi di protezione individuale e di tutti i temi che conosciamo e che abbiamo affrontato. Oggi il Parlamento dà un segnale; è un segnale debole, però è un segnale. Nell'auspicio che tutto questo possa essere l'inizio di un percorso - lo dico anche alla Presidente della nostra Commissione, alla quale ho già avuto modo di formulare i migliori auspici di buon lavoro - il Gruppo Fratelli d'Italia

anche stamattina, nel voto degli articoli, si è riscontrata l'unanimità. Si tratta di un provvedimento di iniziativa del precedente Governo, imposto soprattutto dal moltiplicarsi di episodi di violenza nei confronti dei professionisti sanitari e socio-sanitari.

di aggressioni e violenze, che è l'aspetto più importante e interessante. Per affrontare questo tema abbiamo bisogno di informazione, formazione e comunicazione:

l'articolo 3 pone il tema della promozione dell'informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale sanitario e socio-sanitario, attraverso progetti di comunicazione istituzionale, che dovrà fare il Ministero, e la prevenzione dei protocolli con le Forze di polizia. Si istituisce una giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, attraverso corsi di formazione per il personale medico, una formazione finalizzata alla prevenzione e alla gestione di situazioni di conflitto: dobbiamo formare il nostro personale medico e socio-sanitario e prepararlo a gestire i conflitti, migliorando la qualità della comunicazione tra operatore e cittadini e cittadine utenti. Penso che questi articoli di legge siano essenziali e fondamentali per aggredire questo importante l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, che viene chiamato a collaborare con l'altro Osservatorio nazionale, quello per le buone pratiche sulla sicurezza

pensiamo agli assistenti sociali impegnati nelle periferie delle grandi città, ma non solo, dove c'è una criminalità organizzata molto forte e quanto siano impegnati per aiutare i più deboli.

dei cittadini e delle cittadine si possono riversare su chi è il nostro volto, il volto istituzionale, il volto professionale

per mettere in sicurezza il lavoro di questi professionisti. Ci saranno altri provvedimenti e arriveranno fondi europei. Dobbiamo mettere al primo posto la sicurezza degli operatori,

come neoeletta presidente della Commissione sanità, mi sono recata domenica a Brescia agli Spedali civili ho toccato con mano quanto sia stato fondamentale il lavoro svolto e le condizioni in cui hanno lavorato medici e operatori sanitari delle strutture Dobbiamo fare in modo che questo non avvenga più, dobbiamo sostenerli. C'è una frase che mi hanno detto domenica, che mi ha toccata per cui ho piacere di condividerla in quest'Assemblea. Molti di loro hanno detto di aver lavorato in condizioni di emergenza, senza limiti di orario, senza stare attenti ai turni, insieme, come fossero una comunità: il medico imparava dalle infermiere, le infermiere dal medico, medici di varie specializzazioni condividevano le loro esperienze in quei giorni

la normalità della sicurezza degli operatori sanitari e socio-sanitari. Molti di loro ci dicono di non voler essere considerati eroi, hanno fatto tanto per il nostro Paese e continueranno a farlo, ma noi dobbiamo garantire loro la normalità. Per queste ragioni, in rappresentanza del mio Gruppo Italia Viva-Partito Socialista, voteremo convintamente a favore del provvedimento.

che, come è stato già detto da alcuni colleghi, evidenzia - cercando di dare un segnale - un problema che sta diventando sempre più serio. Bene l'intervento per aggravare le pene in relazione ai reati, bene la prevenzione. Condivido altresì una sottolineatura che faceva il senatore Zaffini. Il provvedimento è stato migliorato alla Camera, ma, oltre al problema della videosorveglianza e dell'aggravamento dei reati, dobbiamo essere consapevoli che, là dell'informazione e della prevenzione, abbiamo un problema di organizzazione delle attività. Voglio fare qualche esempio. I pronto soccorso così non reggono più e creano una situazione di tensione. Ci vuole un intervento di riorganizzazione che preveda percorsi separati, e non dal punto di vista Covid, per chi ha i codici bianchi e per chi, invece, ha situazioni di maggiore gravità.

un aggravamento della situazione dal punto di vista della salute mentale. Stiamo parlando di servizi dove uno o due psichiatri

che affronti in primo luogo anche questi problemi. Solo così potremo dare atto dello sforzo che hanno fatto gli operatori sanitari e socio-sanitari, che non sono eroi: è stato già citato Brecht e non abbiamo bisogno di eroi. Dobbiamo invece rivedere i contratti, dobbiamo dare una soluzione strategica all'assetto organizzativo delle professioni, dobbiamo mettere in discussione le rendite di posizione e dobbiamo riconoscere funzione strategica a professioni che spesso non vedono riconosciuto il proprio ruolo sociale. un ragionamento più generale, vorrei dire culturale. Abbiamo pagato un prezzo, colleghe e colleghi, troppo alto alla narrazione del servizio pubblico come inefficienza e fannulloneria. Ci hanno dimostrato che non è così. Dobbiamo impostare un'altra narrazione in relazione al valore sociale dell'impegno e del servizio pubblico

e non sono solo quelle relative ad una gestione non trasparente del rapporto tra politica e incarichi nella sanità,

Cominciamo a farle perché il nostro servizio ha bisogno di un colpo di reni. i nostri ultimi mesi sono stati sconvolti da un'emergenza sanitaria, la più drammatica dal Dopoguerra, che ha messo a dura prova il nostro sistema sanitario. In questi momenti durissimi il Paese si è stretto in più occasioni, con empatia e gratitudine, attorno al personale sanitario, dai medici agli infermieri che con abnegazione ammirevole hanno affrontato uno tsunami senza precedenti. Alcuni di loro hanno pagato con la loro stessa vita e a tutti va la nostra riconoscenza. In questi mesi difficili è forse possibile rinnovare anche l'alleanza terapeutica fatta di fiducia e rispetto tra medici, *équipe* e pazienti. Una relazione che si fonda sulla presa in carico del malato con le sue paure e con le sue fragilità. Prima che si scatenasse questa drammatica epidemia, si stava diffondendo un crescendo di aggressioni contro il personale sanitario un'alleanza si stava spezzando tra insulti, intimidazioni, aggressioni fisiche e verbali. Sui giornali abbiamo letto di notti da incubo tra urla, minacce e violenze, che si consumavano in qualche pronto soccorso. Si parlava letteralmente di medici sotto assedio, un problema drammatico perché, come purtroppo abbiamo appreso in questi ultimi mesi, l'esperienza sanitaria e l'assistenza, la cura dei malati, riguarda tutta la società e ha un ruolo essenziale. La sua tenuta passa dalla valorizzazione delle risorse, delle donne e degli uomini che ne costituiscono la spina dorsale e che devono poter lavorare in sicurezza. In un momento storico come questo, in cui sono sempre più forti le tensioni sociali, non possono sfibrarsi proprio i rapporti su cui si costruiscono le nostre comunità. Le aggressioni contro il personale sanitario sono particolarmente inquietanti perché si tratta di violenze contro chi si prende cura di noi nei momenti fragili della malattia. Secondo un'analisi dell'Anaao-Assomed, il 65 per cento dei medici dichiara di essere stato vittima di aggressioni fisiche o verbali. Questa percentuale impressionante sale all'80 per i medici in servizio al pronto soccorso o al 118. Nel 2019 i numeri ufficiali parlavano di oltre 1.000 episodi, senza tener conto delle aggressioni non denunciate, che ci porterebbero a triplicare questi numeri. una vera e propria emergenza, che coinvolge persone che svolgono attività di cura in contesti emotivamente, oltre che sanitariamente, complessi e che proprio per questo devono essere maggiormente tutelate. Non ci sono giustificazioni a queste violenze, bisogna condannare queste condotte, prima e dopo la pandemia. In tal senso, il provvedimento in esame, che conclude oggi il suo *iter* parlamentare, non è soltanto giusto, ma necessario. Sarà finalmente applicata l'estensione delle stesse pene previste nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a pubblico ufficiale, anche al personale delle professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle proprie funzioni. A ciò si aggiunga che queste professioni saranno tutelate, prevedendo un'ulteriore aggravante per chi commette il fatto con violenza o minaccia, proprio in ragione della professione di chi la subisce. giusto, inoltre, l'aggravio delle pene in caso di lesioni gravi o gravissime, anche a danno di «chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso». Un ringraziamento va quindi ai colleghi deputati, che nell'ambito del passaggio parlamentare alla Camera hanno rafforzato e implementato alcuni ulteriori e importanti misure in tal senso. Colleghi, non basta però inasprire le pene, se non si agisce anche a livello culturale e organizzativo del sistema sanitario, anche attraverso una migliore organizzazione dei turni di lavoro una formazione alla relazione e alla gestione della propria vita emotiva, all'adozione di princìpi specifici nei protocolli di sicurezza, alla promozione del lavoro di *équipe*. Non si deve dimenticare, infatti, che l'esposizione prolungata al dolore, nelle professioni mediche è fonte, notoriamente, di grande *burnout* e di difficoltà emotive anche forti, al punto che la letteratura scientifica parla persino di un tasso suicidario più elevato nei medici. Ben venga quindi il provvedimento, che cerca di dare risposte, anche con la promozione di iniziative di formazione e informazione sull'importanza del rispetto del lavoro sanitario, attraverso la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale, la prevenzione delle situazioni di conflitto l'istituzione di una giornata di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura nuova, attraverso una maggiore informazione e formazione. È importante sottolineare che non esistono relazioni di cura prive di emozioni: è l'atteggiamento di chi ostenta freddezza emotiva, che spesso maschera, sotto l'apparente impassibilità, una difesa davanti al continuo contatto con la sofferenza. In fondo, già la mitologia greca ci raccontava del centauro Chirone, il guaritore ferito, ferito, colpito da una freccia che gli aveva procurato una ferita inguaribile, che ogni giorno, prima di andare ad insegnare l'arte medica agli altri, doveva curare se stesso: curare e prendersi cura di sé, per poter prendersi cura degli altri. Le professioni sanitarie sono complesse e difficili e spesso il personale non è adeguatamente preparato a riconoscere le proprie emozioni, ma anche a gestire o contenere l'aggressività dei pazienti o delle loro famiglie, che magari non accettano il dolore di una diagnosi infausta grazie a tutti una preparazione, che solo raramente entra a far parte del bagaglio formativo delle professioni sanitarie. Sia chiaro allora che, se da una parte sono certamente comprensibili, in certi casi, la protesta e la richiesta di attenzione e responsabilizzazione nei confronti di possibili errori o di migliorare la comunicazione, dall'altra non è accettabile che l'esercizio della professione medica sia oggetto di aggressione, ostacolata da eccessi drammatici e ingiustificati. Non dimentichiamo che la relazione tra malato e medico è relazione tra chi sta male e chi può guarirlo, perciò si deve fondare su fiducia e rispetto reciproco. Speriamo che questi mesi di grande dolore ci abbiano dato l'opportunità di riscoprire e di rinsaldare un patto;

Occorre dunque rileggere con sguardo nuovo, con occhi nuovi, lo stesso percorso formativo sanitario, ponendo al centro della relazione di cura le persone che, nella loro unicità, non possono essere incasellate, classificate, ridotte a organi, perché stiamo parlando di corpi-persona. In una prospettiva di umanizzazione dei servizi è quindi necessario potenziare il prendersi cura di chi si prende cura (lo ripeto: prendersi cura di chi si prende cura), per un agire professionale fatto certamente di abilità tecnica e di competenza sanitaria, ma anche di saggezza esistenziale.

quando c'è la volontà politica ed istituzionale, si può esprimere la migliore sintesi normativa possibile. Senza polemica alcuna, l'auspicio è che anche su altre tematiche di particolare interesse per i cittadini del nostro Paese, come per esempio l'utilizzo dei fondi europei che sono sicuramente utili per dare un ampio respiro all'economia del nostro Paese, si possa arrivare alla condivisione degli obiettivi e quindi degli strumenti normativi per raggiungere i fini prefissati.

del Gruppo Forza Italia, Anna Maria Bernini - al disegno di legge in esame, che reca importanti disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Lasciatemi rivolgere un pensiero affettuoso e riconoscente ai colleghi medici e al personale paramedico e socio-sanitario che, durante la grave pandemia che ci ha colpiti, hanno dato dimostrazione di grande professionalità, senso del dovere, abnegazione e coraggio. A tutti loro deve pervenire il nostro più accorato Passando all'esame del merito del provvedimento oggi in discussione, l'articolo 2 del disegno di legge prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, che sarà un importante strumento per rilevare le situazioni di maggiore esposizione a rischio del personale medico e paramedico, che spesso purtroppo, oltre a pensare a salvare le vite degli altri, sono in balia di soggetti che commettono atti di violenza nei loro confronti. Il disegno di legge prevede anche la promozione di iniziative volte ad informare sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché l'aggravamento delle pene per i casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate ai nostri professionisti del mondo della sanità. prevede che i reati in danno del personale sanitario divengano perseguibili d'ufficio e non più solo a querela della persona offesa. Particolare importanza riveste anche l'istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. L'attività di prevenzione ed educazione, in tutti i casi di comportamenti socialmente devianti, è la via maestra, molto più importante dell'attività repressiva e sanzionatoria: è fondamentale trasmettere alle nuove generazioni quel senso di rispetto e gratitudine nei confronti di figure fondamentali della nostra società come i docenti e i medici. I nostri padri e i nostri nonni vivevano questo rispetto e questo senso di gratitudine e il prestigio sociale che circondava la figura del medico, come quella del docente, era disancorato dal livello di redditività che oggi appare l'unico parametro di valutazione. Colleghi senatori, onorevoli membri del Governo, Forza Italia ha voluto dare un grande contributo al provvedimento presentando un ordine del giorno che impegna l'Esecutivo a un preciso e dettagliato monitoraggio degli effetti di questo disegno di legge, al fine di modificare e correggere tutto ciò che dovesse dimostrarsi inefficace e inefficiente. In particolare, abbiamo evidenziato nell'ordine del giorno che tra i compiti dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 vi è il monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza. Abbiamo segnalato che la raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari del Ministero della salute intende incoraggiare l'analisi dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati, l'adozione di iniziative e programmi volti a prevenire gli atti di violenza e/o attenuarne le conseguenze negative e, pertanto, l'individuazione delle più adeguate condizioni di sicurezza dei presidi sanitari ospedalieri in quanto luoghi di lavoro (sapete bene cosa accade nei Pronto soccorso del nostro Paese ogni giorno). Deve considerarsi questa la condizione inderogabile al fine di salvaguardare la più sicura operatività del personale, senza trascurare la sicurezza dei pazienti e degli utenti delle strutture sanitarie ospedaliere. La preoccupazione infatti è che, sebbene in queste ultime settimane sia stata attuata una sorta di rivalutazione dell'immagine di medici e infermieri, che sono diventati eroi nazionali e guerrieri in prima linea, il fenomeno della violenza ai danni del personale sanitario sia molto più diffuso e persino in continuo aumento. Il 28 aprile, pochi mesi fa, l'Organizzazione mondiale della sanità, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, ha invitato tutti i Governi, le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, nonché la comunità globale, ad adottare misure urgenti per rafforzare le capacità delle Nazioni di proteggere la salute sul lavoro e la sicurezza degli operatori sanitari. Come sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanità, dall'8 al 38 per cento degli operatori sanitari nel corso della loro carriera subisce violenze fisiche. Il Governo, esprimendo parere favorevole all'ordine del giorno da noi presentato come allegato al provvedimento, si è impegnato a valutare l'opportunità, all'esito del monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti in esame, di prevedere ulteriori misure volte a consentire un più ampio e diffuso utilizzo di strumenti di videosorveglianza nelle strutture sanitarie e negli ambienti individuati dalla legge, così come in ulteriori ambiti, come la sicurezza nelle strutture per l'infanzia, per gli anziani e per persone con disabilità. Si è impegnato inoltre a favorire la conclusione dell'*iter* parlamentare delle proposte di legge volte a prevenire e contrastare condotte di maltrattamento e abuso, anche mediante l'utilizzo di strumenti videosorveglianza. Stanti il lavoro congiunto e l'accoglimento dell'ordine del giorno da noi presentato,

era stato promosso anche dall'allora ministro dell'interno Matteo Salvini. Già dal titolo infatti quali avrebbero dovuto essere gli obiettivi della Lega e di quel Governo di questa legislatura, «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni». Si sa che le dinamiche cambiano. Dopo i risvolti degli ultimi mesi, c'è da chiedersi - legittimamente - se per voi sia chiaro il concetto semantico racchiuso nella parola «sicurezza».

concreta e consapevole di tutela del personale sanitario e socio-sanitario. Ma siete veramente convinti che promuovere le buone prassi e istituire un osservatorio sia veramente sufficiente a proteggere medici, infermieri, operatori sanitari e tutta la filiera sul campo? No, signori, non è sufficiente starsene seduti in un ufficio in compagnia di rappresentanti di organizzazioni sindacali e di categoria e delle Regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti. Durante l'esame in seconda lettura alla Camera dei deputati avete inserito anche l'INPS: con l'aggiunta di un paio di *task force* avremmo potuto dire che sareste state delle personcine veramente - prevede l'istituzione della "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari", Bello! Ma secondo voi una giornata sul calendario è un aiuto concreto per chi si prende schiaffi, sputi, coltellate, stupri e spari? Parlo naturalmente dei Pronto soccorso e dei centri di salute mentale, che oggi sono ancora un tabù di cui nessuno ha iniziato a parlare. Questo Governo ha una strana maniera di intendere la sicurezza con il provvedimento in esame: da una parte, ad aggressione avvenuta e crimine commesso, si tutela obbligando le aziende sanitarie a costituirsi parte civile; dall'altra, si respingono però gli emendamenti che richiedevano la videosorveglianza e un presidio fisso di polizia, anche con un solo agente, non tanto per essere pronti a intervenire in caso di emergenza, ma per

100 miliardi di euro, nessuno ha pensato di rivedere la propria posizione a favore e doverosa tutela del personale sanitario e socio-sanitario? Non vi sarebbe caduta la corona di latta. Eppure, sono già stati stanziati 30 milioni di euro per anno, dal 2020 al 2024. Sembrerebbe che, per voi, la priorità siano gli osservatori, le buone prassi, le giornate del ricordo e la promozione dell'informazione. In sostanza, un giro di valzer; ma siete al Governo e vi siete anche circondati di un esercito di altre 450 persone! Voteremo sì, perché auspichiamo che questo sia solo il preludio di una presa in carico sincera. Ora che siamo stati stravolti dall'esperienza Covid-19 e che siamo sopravvissuti alla stessa, ora che siamo ancora più consapevoli, questo atto non può essere il massimo che l'attuale Governo può offrire a medici, infermieri e operatori, perché, così com'è, quest'atto non è neanche il minimo.

oggi abbiamo il dovere di consegnare finalmente al Paese un provvedimento di civiltà non più procrastinabile. Mi sono impegnata in prima persona affinché si accelerasse l'*iter* conclusivo di questo disegno di legge, che ha un forte valore sociale e rappresenta un preciso dovere politico a salvaguardia dell'incolumità di chi tutela le nostre vite e tutela quel diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Quello delle aggressioni al personale sanitario è ormai un fenomeno di portata preoccupante, una vera e propria emergenza se pensiamo che ogni anno vengono denunciate circa 1.400 aggressioni: quasi quattro al giorno. di dati parziali, perché spesso gli operatori sono reticenti a portare alla luce inadeguatezze strutturali o a interrompere il turno di lavoro o persino a causare danno agli aggressori. Gli episodi reali sono molti di più: si stima, infatti, che siano oltre tremila i casi di aggressioni a medici e infermieri in un anno. Oltre alle aggressioni fisiche, vanno considerati anche tutti i comportamenti lesivi della dignità dei professionisti sanitari, comprensivi di insulti e minacce; comportamenti che non possono essere sottovalutati. La concentrazione più alta di questi casi si registra nel Mezzogiorno, con il 72 per cento al Sud e nelle isole. Per l'80 per cento, queste aggressioni interessano il personale impegnato nei reparti di emergenza e urgenza, sia ospedaliera che territoriale, perlopiù in strutture pubbliche; ennesima prova, questa, del profondo divario interregionale determinato da politiche inadeguate, che hanno smantellato le reti territoriali che dovevano fare da filtro. Si pensi che al Sud, negli ultimi anni, sono stati chiusi 42 piccoli centri ospedalieri. Politiche che hanno generato il sovraffollamento dei nostri nosocomi. e quindi dei Pronto soccorso, e hanno trasformato le osservazioni intensive brevi in veri e propri reparti di degenza. Chi lavora per salvare vite umane non può farlo in condizioni di pericolo della propria incolumità; condizioni create da anni di tagli, che hanno prodotto lunghe liste d'attesa e prese in carico tardive e poco adeguate, che spesso sono causa di esasperazione degli utenti. Tagli impietosi, che hanno falciato diritti e possibilità, avvenuti in un settore fondamentale per il benessere di un Paese, nel quale non bisognerebbe mai smettere di investire e che dovrebbe essere una priorità per tutte le forze politiche, inclusa quella cui appartengo. L'emergenza Covid-19 ha mostrato ancora di più, semmai ve ne fosse bisogno, quanto le risorse umane siano determinanti per la tenuta del Servizio sanitario nazionale. Abbiamo chiamato gli operatori «eroi», abbiamo dedicato loro parole emozionanti, abbiamo ristabilito con loro un rapporto di fiducia perché è risultato evidente che, grazie a tutti loro, sono state salvate migliaia di vite. Adesso, però, dobbiamo loro atti concreti e non più solo promesse, perché chi salva vite umane non deve rischiare la propria. Questo è un paradosso moralmente inaccettabile. A tal proposito, vorrei sollecitare tutti i miei colleghi di maggioranza e di opposizione a riprendere al più presto la discussione sullo scudo legale per i medici che hanno operato nelle corsie durante i mesi più difficili dell'emergenza Covid. discussione si è arenata perché molti, oltre a tutelare il personale in trincea, hanno provato a mettere uno scudo anche alle dirigenze, che invece, a nostro avviso, devono assumersi la responsabilità della mancata programmazione a gestire l'emergenza e del non aver saputo mettere al sicuro innanzitutto il proprio personale. Questa legge contro le aggressioni in sanità, fortemente voluta dall'*ex* ministro alla salute Giulia Grillo, è stata oggetto di un lungo lavoro in Commissione sanità al Senato, dove sono state inserite importanti modifiche, tra cui la procedibilità d'ufficio. Abbiamo lavorato senza sosta coinvolgendo tutti gli attori in campo attraverso un lungo ciclo di audizioni che ha portato all'integrazione del testo base con misure ritenute essenziali dagli stessi operatori sanitari, tra cui, ad esempio, le modifiche al codice penale che estendono a tutti i casi di aggressioni al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria le pene aggravate previste per le corrispondenti ipotesi di lesioni cagionate a un pubblico ufficiale prevedendo sempre, come dicevo, la procedibilità d'ufficio e senza la necessità che vi sia querela da parte della persona rispondo anche al senatore Zaffini perché in questo modo abbiamo previsto un trattamento equiparabile a quello riservato a un pubblico ufficiale recependo l'indirizzo della Corte di cassazione, che stabilisce lo stato di pubblico ufficiale non con riferimento all'intera funzione devoluta devoluta dalla legge, bensì con riguardo ai singoli momenti in cui l'attività stessa viene concretamente esercitata. In questo modo, gli operatori sanitari beneficeranno di tutte le tutele previste per i pubblici ufficiali, ma senza averne gli oneri. Sarà, inoltre, preziosa l'istituzione dell'Osservatorio sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie grazie alla quale sarà possibile non solo monitorare gli episodi di violenza, ma anche promuovere studi e analisi per poter porre in essere misure per poter porre in essere misure idonee alla rimozione dei fattori di rischio negli ambienti più esposti. Alla Camera era stato introdotto in Commissione l'obbligo di costituzione di parte civile da parte delle ASL e degli ospedali, che a mio avviso era un'aggiunta importante, ma poi con un emendamento soppressivo dell'opposizione in Aula si è tornati al testo precedente. Altro punto cruciale in questa legge è la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria. Questo è un aspetto fondamentale perché per costruire una nuova visione è sempre necessario anche un cambiamento culturale e di questa nuova visione i cittadini devono essere parte attiva e consapevole. Ad esempio, mi piace pensare che, responsabilmente e grazie al coinvolgimento e all'informazione corretta, tutti i cittadini prendano coscienza che usare la mascherina e rispettare il distanziamento serve anche a evitare che quelli che chiamiamo eroi debbano di nuovo indossare gli "scafandri" e portare sul viso i lividi e i segni i segni del dolore e della fatica al limite della sopportazione. (*Applausi*). Chiaramente non basterà una legge a tessere una solida rete di protezione intorno al nostro personale sanitario, ma bisogna impegnarsi a costruire quella alleanza tra medico e paziente che una volta era salda e che poi è stata inficiata dai tagli, dai pochi mezzi della sanità pubblica e da chi non ha perso occasione per far ricadere proprio sugli operatori ogni responsabilità, senza capire che il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale deve partire innanzitutto dalla revisione dei criteri di nomina dei dirigenti. Se in un'azienda o in un ospedale non sono stati costruiti percorsi di accesso adatti, non si è saputo incidere sulle liste di attesa, non sono state fornite ai propri dipendenti tutte le armi necessarie per assistere i pazienti nel modo migliore, allora la responsabilità è di chi non ha saputo programmare. Non ci si improvvisa esperti di sanità, non basta un corso regionale di poche ore per garantire l'accesso all'elenco dei direttori generali: questa non è meritocrazia, ma è mortificazione del merito per salvare l'appartenenza e la fede politica. All'inizio di questa legislatura ho depositato un disegno di legge che rivede proprio i criteri di nomina dei direttori generali, amministrativi e sanitari per garantire che a capo di ASL ed ospedali ci siano i più esperti e i più capaci. Quel disegno di legge è ancora fermo in Commissione ed oggi sollecito il Governo a farsi carico di questa riforma, impegnandosi a garantire il presupposto per fornire alle nostre eccellenze tutti gli strumenti e le condizioni per poter svolgere al meglio il loro delicato compito. Dobbiamo lottare per eliminare l'ingerenza politica nel sistema delle nomine. Dobbiamo rivedere il percorso di formazione dei medici. Anche su questa riforma, incardinata in Commissione, sono certa che i miei colleghi abbiano il mio stesso interesse ad approvarla in tempi rapidi. Dobbiamo rafforzare la medicina territoriale, rivoluzionare l'emergenza-urgenza, livellare i divari regionali, puntare su una sanità pubblica di qualità e con una sanità privata che faccia da stampella... che assorbe risorse senza erogare i servizi. Il voto favorevole che oggi esprimo, a nome del mio Gruppo MoVimento 5 Stelle, deriva dalla consapevolezza che sarà soprattutto questo impegno e questa visione a proteggere il diritto alla salute previsto dalla nostra Carta costituzionale e a permettere al nostro Servizio sanitario nazionale di saper affrontare le sfide che verranno, partendo proprio dalla tutela e dalla valorizzazione di tutto il personale.

Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto tra l'Italia e l'Argentina nel settembre 2016. L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato dalle Camere, risponde all'esigenza di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza. Il testo, che si compone di un preambolo e di 12 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'intesa (articolo 1), individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare all'elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed all'organizzazione di visite reciproche di delegazioni e di scambi di esperienze tra esperti, nonché la partecipazione a corsi di esercitazione (articolo 2). Tra i campi di cooperazione sono annoverati i settori della sicurezza comune e della politica di difesa, della ricerca e sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa,

si compone di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li quantifica in 5.504 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020 imputabili alle sole spese di missione. L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Grazie, Presidente. l'Accordo la cui ratifica stiamo trattando, così come istituito, ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. I suoi obiettivi e le sue finalità sono condivisibili, in quanto mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi. Infatti i suoi princìpi ispiratori intendono incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei princìpi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle parti, nel pieno rispetto delle relative organizzazioni sovranazionali e in particolare, per la parte italiana, dell'ordinamento dell'Unione europea e, per la parte argentina, dell'Unione delle Nazioni sudamericane. Con tale Accordo si cristallizzano i campi di maggiore interesse della costituita cooperazione, tra i quali si evidenziano i settori della sicurezza comune e della politica di difesa, la ricerca, lo sviluppo e l'acquisizione di prodotti e servizi per la difesa. Si è poi inciso sui campi della partecipazione a operazioni di mantenimento della pace e umanitarie internazionali, nonché su formazione, istruzione ed esercitazioni militari. Punti favorevoli di tale Accordo si riscontrano anche nelle disposizioni che disciplinano gli aspetti attinenti alla giurisdizione sul personale ospitato nei rispettivi Paesi, alla protezione della proprietà intellettuale, alla sicurezza dell'informazione e alla risoluzione delle controversie, la cui disciplina viene sempre imperniata sul principio della leale cooperazione tra i Paesi interessati e nel pieno rispetto, sia dal punto di vista della legittimità che della compatibilità, delle norme e dell'ordinamento dell'Unione europea. Tale visione di cooperazione si inserisce in modo compatibile con la strategia globale per la politica estera, tesa a un'effettiva difesa comune dell'Unione europea attraverso la collaborazione permanente tra gli Stati membri impegnati. È per tali motivi che Fratelli d'Italia è favorevole alla ratifica di tale Accordo, che contribuisce a mantenere sempre più coesi i rapporti tra i due Paesi, storicamente legati da comuni principi e valori cristiani. Pertanto auspichiamo che la stessa rappresenti la naturale continuazione di un rapporto bilaterale oramai consolidatosi negli anni, tanto da rappresentare una visibile e significativa realtà di cooperazione tra i due Paesi.

Mi permetta comunque di sottolineare solamente un piccolo aspetto: fra l'Italia e l'Argentina c'è una collaborazione continua e si crede in valori

Anche per queste ragioni, penso che questa ratifica non faccia che accrescere e sostanziare la vicinanza tra i due Paesi. Il Gruppo Partito Democratico voterà pertanto a favore della ratifica di questo Accordo.

ci apprestiamo a ratificare sancisce un Accordo di cooperazione tra l'Italia e l'Argentina in ambito militare ed ha come fine ultimo quello di stringere la cooperazione militare tra i due Paesi. Tali ratifiche sono estremamente importanti per diversi motivi. Prima di tutto, possono servire da volano nel provocare effetti indiretti dal punto di vista commerciale, in quanto riguardano un settore, come quello militare,

ma lo stesso si può dire per le altre tipologie di accordo di cooperazione bilaterale - forniscono all'Italia un importantissimo strumento di diplomazia, che rischia invece di venire oscurato in contesti multilaterali. L'Italia nell'ambito della cooperazione, privata o pubblica che sia, rimane un'eccellenza. Tali accordi vanno incentivati e intensificati, onde ripristinare l'immagine dell'interesse dell'Italia sul piano internazionale, tanto più in una regione strategica per noi e per la nostra diplomazia come quella latino-americana. Non scordiamoci dei tantissimi cittadini italiani presenti in America latina: parliamo di circa un milione di persone,

Pensiamo solamente al grido di aiuto che la nostra comunità italiana in Venezuela continua a rivolgerci e che troppo spesso è rimasto inascoltato. Come ho detto, la regione latino-americana è importante, ma ancora più importante è il rapporto con l'Argentina. Pensate che in questo Paese è presente una comunità di cittadini italiani che sfiora un milione di persone: una Regione italiana aggiuntiva. È fondamentale che in contesti come questi l'Italia sfrutti appieno le sue capacità di *soft power* nell'ambito culturale in quello militare, passando per gli sbocchi commerciali che mai come oggi abbiamo tanto bisogno di intensificare, dopo la crisi economica causata dalla crisi sanitaria, che ha investito maggiormente anche il nostro Paese. Avere *partner* forti e sinergie affidabili in tutti i contesti regionali deve essere una prerogativa per il nostro Paese e l'Italia ha tutte le carte per perseguire tale scopo.

Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, l'Accordo in esame intende incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dell'Italia e dell'Argentina per consolidare le rispettive capacità

oltre 900.000 cittadini italiani vivono oggi in Argentina, una comunità alla quale dobbiamo molto e alla quale, ripeto, siamo molto legati. Al momento della sua entrata in vigore, questo Accordo sostituirà quello di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dai due Paesi a Roma il 6 ottobre 1992 e ratificato dall'Italia con la legge n. 173 del 1996, entrato poi in vigore il 21 luglio 1997. I settori della cooperazione bilaterale si riferiscono all'elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali, all'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienza tra esperti e alla partecipazione a corsi ed esercitazioni militari. In particolare, i campi di cooperazione attengono a: sicurezza comune e politica di difesa; ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; proprietà intellettuale e brevetti; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; organizzazione e impiego delle Forze Armate, nonché strutture ed equipaggiamento di unità militari e gestione del personale; formazione e addestramento in campo militare; sanità militare e sport militare. Infine, voglio ricordare che, con l'abolizione (nel 2008) del codice di giustizia militare, l'Argentina - già abolizionista, nel 1984, per i crimini ordinari - ha cancellato definitivamente la pena di morte dal proprio ordinamento. L'accordo, oltre a rafforzare il legame tra il nostro Paese e l'Argentina, costituisce, dunque, un'intensa un'intensa attività intergovernativa idonea a semplificare la procedura di autorizzazione alle trattative contrattuali e all'esportazione e importazione di materiale d'armamento, fatti salvi i divieti imposti dalla legge n. 185 del 1990. Per tutte queste ragioni, esprimo il voto favorevole di Forza Italia, notando che, finalmente, tutta l'Assemblea si rende conto dell'importanza di stabilire rapporti anche in tema di armamenti. È vero che c'è una conversione importante anche da parte di certi settori - non me lo sarei mai aspettato - che finalmente cominciano a comprendere che, se vogliamo realizzare la pace, dobbiamo anche arrivare a una difesa armata. Diceva la saggezza latina - non ce ne dobbiamo dimenticare - *si vis pacem, para bellum*. Per queste ragioni, il Gruppo Forza Italia voterà favorevolmente al disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo.

tra Italia e Argentina affonda le sue radici nella presenza di tanti nostri connazionali in quel Paese e, anche se a volte si mette in discussione la limpidezza di questo rapporto, essa appare sempre più nel suo fulgore. Consentitemi di dire che, nei mesi scorsi, la neo eletta vice presidente della Repubblica, la signora Kirchner, ha detto cose assai sgradevoli dell'Italia;

questo sentimento è stato suffragato da un incontro ufficiale - proprio all'indomani di quell'affermazione - con l'ottimo ambasciatore italiano Manzo. Credo che questa occasione, per quanto mi riguarda, debba coincidere con l'affermare i sentimenti di amicizia e di vicinanza al popolo argentino, che in questo momento, anche per via della stagione invernale,

tra la Repubblica italiana e quella argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016. Un medesimo disegno di legge di ratifica era già stato esaminato nel dicembre 2017 dalla Commissione esteri del Senato con atto n. 2969, ma l'esame non poté la sua conclusione perché finì la XVII legislatura. L'accordo in esame ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato e risponde all'esigenza di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate di Italia e Argentina con il preciso intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza. Il testo bilaterale, come è stato ben illustrato dalla relatrice, si compone di un preambolo e di 12 articoli; dopo aver enunciato princìpi e scopi di intesa, individua le modalità attuative e i settori della cooperazione, riferendosi in particolare all'elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali, all'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, a scambi di esperienze tra esperti e partecipazione a corsi ed esercitazioni militari. È quindi di fondamentale importanza sottolineare come tra i campi di cooperazione siano annoverati i settori della sicurezza comune, della politica di difesa, della ricerca, dello sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni di mantenimento della pace con il supporto delle Nazioni Unite, dell'organizzazione ed impiego di Forze armate, della formazione delle stesse e della sanità militare. È chiaro quindi che il testo identifica le categorie di materiali della Difesa interessate da una possibile collaborazione bilaterale, prevedendo l'impegno delle parti a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito senza il preventivo benestare della parte cedente. Se è vero, dunque, che l'accordo in questione ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale, non può però passare in secondo piano che la sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche ad indurre effetti positivi ed effetti indiretti in diversi settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

legami unici imprenditoriali che è impossibile non tenere in considerazione, a partire dal fenomeno della storica emigrazione italiana verso il territorio dell'attuale Repubblica Argentina, passando attraverso il commercio bilaterale che, oltre ad essere concentrato su prodotti di generi alimentari, riguarda anche macchinari e strumentazioni scientifiche di vario tipo. L'Italia è dunque un investitore di rilievo in Argentina e quando il Governo Conte si è insediato, in tanti si sono chiesti quale atteggiamento avrebbe assunto nei confronti della difesa del nostro Paese, in numerosi si sono preoccupati o addirittura hanno inteso speculare sui dubbi da instillare, su come il MoVimento 5 Stelle, per via del forte legame con il suo elettorato, avrebbe affrontato i temi legati alle Forze armate. Ebbene, in tanti si sono dovuti ricredere. Eliminare le spese inutili in ogni campo, Difesa compresa, è e rimane per il MoVimento 5 Stelle una stella polare, ma la *leadership* è consapevole degli equilibri internazionali e della necessità della difesa del Paese, da valorizzare ed incentivare nella giusta misura. misura. Rimando quindi all'importanza dell'articolo 6, che elenca proprio i materiali per la difesa che possono essere oggetto di cooperazione, fermo restando il rispetto delle legislazioni nazionali di entrambi i Paesi. Ricordo, per l'Italia, la legge del 9 luglio 1990, la n. 185, sulle esportazioni di materiali d'armamento al pari del divieto di esportazione del materiale acquisito che è di fondamentale e dirimente importanza. Prima di annunciare il voto del Gruppo MoVimento 5 Stelle, a proposito di cooperazione, non posso fare a meno di aprire uno spaccato - e prego l'Assemblea di fare attenzione di fare attenzione - su quanto è accaduto ieri a Beirut. Il Libano è stato dilaniato ancora una volta da due forti esplosioni che hanno portato a tantissimi feriti e soprattutto al ferimento di due soldati italiani della Marina militare ai quali noi, come Gruppo MoVimento 5 Stelle, vogliamo portare la nostra solidarietà e il nostro augurio di pronta guarigione. Approfitto ancora di pochi secondi per fare nostre, mie, le parole del ministro Di Maio: «l'Italia è vicina agli amici libanesi in questo momento tragico. I nostri pensieri vanno alle famiglie delle vittime a cui esprimiamo il nostro profondo cordoglio, e alle persone ferite a cui auguriamo una pronta guarigione». Aggiungo da parte nostra un abbraccio forte e grande per tutto il contingente italiano impegnato in Libano.

ha appena contattato i Capigruppo, dicendo che il Governo si è accorto, ahimè in modo un po' tardivo, che il 10 agosto scade il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e quindi, per legge, bisogna venire in Assemblea con le comunicazioni e rispettare il fatto che prima venga data informativa a tutta l'Assemblea. bisogna venire in Assemblea a fare il proprio dovere, rispettando la legge. Questo è quanto deve essere fatto: la seduta fino alle ore 15, che riprenderà con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione.

Presidente, la ringrazio per

dare moltissimo alla sua terra e alla comunità nella quale è vissuto. Bruno Dettori, sassarese, era un docente universitario della prestigiosa facoltà di agraria dell'Università degli (con un breve intervallo, nel quale ha insegnato all'università in Eritrea). È stato autore di innumerevoli pubblicazioni su riviste, nazionali e internazionali, di idrogeologia, idrochimica e approvvigionamento idrico. una brillante carriera professionale, che non gli ha impedito però di coltivare la sua profonda passione per la politica, nella quale ha fatto la gavetta, essendo stato consigliere comunale e regionale, senatore e Sottosegretario all'ambiente nella legislatura 2006-2008 col Governo Prodi. Questo è stato il suo brillante *curriculum* dell'attività politica, ma di Bruno Dettori credo sia più giusto ricordare il tratto umano, che lo ha condotto a diventare un importante punto di riferimento per tutti coloro che l'hanno conosciuto o hanno avuto il piacere di collaborare con lui. Con una modestia e umiltà fuori dal comune, ha sempre manifestato capacità di ascolto nei confronti di chiunque volesse parlare con lui, anche i più deboli e le categorie ingiustamente considerate ultime. A tutti elargiva un consiglio e manifestava vicinanza e considerazione, prodigandosi nella ricerca della soluzione ai loro problemi. Non posso non ricordare una caratteristica fondamentale di Bruno Dettori, del quale sono stato amico per parecchi anni. anni. Una volta lasciati i ruoli istituzionali, egli ha assunto la veste di padre nobile nell'ambito del suo partito, continuando a coltivare quella passione per la politica che ha connotato la sua vita e l'attività a favore della collettività, prodigandosi per il ricambio generazionale. Questa è stata una caratteristica importantissima, grazie alla quale ha aiutato molti giovani ad emergere nella vita politica, così favorendo, come dicevo, il ricambio generazionale della classe politica. Egli si è sempre prodigato per cercare di risolvere i conflitti interni al partito, ma anche i contrasti con le altre forze politiche. Ha fatto ciò con una ricerca continua del dialogo continua del dialogo con tutti. Anche nei momenti più difficili non è mancata una sua telefonata di sostegno e stimolo a reggere il confronto. Chi ha avuto il piacere di conoscerlo non potrà dimenticare il suo sorriso sincero, aperto e accattivante, il suo ottimismo contagioso e stimolante e la sua profonda umanità. A nome di tutto il Gruppo Italia Viva, esprimo cordoglio, rimpianto e vicinanza alla signora Isa, il mio intervento si muove in continuità con quello del collega Cucca, con una piccola differenza, perché io ho avuto modo di collaborare con il consigliere regionale Bruno Dettori dal 1994 al 2001: anni di particolare intensità politica, durante i quali, pur militando su fronti diversi, si riusciva a trovare con lui una sintesi sui progetti che potevano risultare qualificanti per l'isola.

Mi dispiace veramente dover fare le condoglianze alla famiglia, perché la Sardegna ha certamente perso un punto di riferimento nella politica. Infatti, terminato il suo impegno diretto

Nell'esprimere il cordoglio di Forza Italia a tutta la famiglia, ne ricordiamo la figura e sono sicuro che non solo Sassari sentirà la sua mancanza. *(Applausi)*. Ringrazio il senatore Cucca e il senatore Floris per questo ricordo, cui unisco il mio cordoglio. Avendo avuto la fortuna di averlo conosciuto personalmente, non posso dimenticare il suo saper essere una persona perbene e l'amore che aveva per la sua terra, la Sardegna. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Torino, VI sezione penale. Con ricorso, depositato il 20 febbraio 2020, il tribunale ordinario di Torino, VI sezione penale, ha sollevato un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti del nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 9 gennaio 2019, ha dichiarato l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni rese da Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi allo stesso tribunale ordinario di Torino. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale, con l'ordinanza del 26 maggio 2020, n. 148, depositata in cancelleria il successivo 10 luglio 2020. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 30 luglio 2020. Nella seduta del 4 agosto 2020 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso a maggioranza parere favorevole alla costituzione

ha proposto di sostenere la decisione di costituirsi in giudizio per difendere la deliberazione del Senato. Ricordo a me stesso che è la prassi che generalmente il Senato segue. Pertanto, in rappresentanza della maggioranza

Signor Presidente, impiegherò molto meno tempo di quello che lei mi ha concesso per dire che il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore della proposta del presidente Gasparri. Credo che il Senato non solo abbia il diritto, ma abbia anche il dovere di difendere le proprie deliberazioni, qualora si renda necessario, nel caso in cui, come in questa circostanza, vengono contestate con un conflitto di attribuzione

la dichiarazione di voto di oggi potrebbe iniziare e finire con due assunti: si tratta di una decisione votata all'unanimità dalla Giunta come giustamente ha detto il collega che mi ha preceduto, il Senato è tenuto istituzionalmente a difendere le proprie deliberazioni.

Abbiamo avuto diverse occasioni di discussione in quest'Aula di tutto ciò che ha a che vedere con le prerogative del Parlamento, dei suoi componenti e del Governo nel rapporto con gli altri poteri dello Stato e, quindi, con la

parlamentare o membro di un Governo uno *status*. Quando prendiamo queste decisioni, compresa quella di oggi, non stiamo difendendo uno *status* di ottimati o

è a difesa della funzione del parlamentare e, quindi, la libertà del parlamentare è a difesa di questo genere di attività. Per questo possiamo,

di quei poteri che, nella fattispecie, ci vedono in un rapporto di contrapposizione dialettica di chi rivendica un'esclusiva. può sembrare superflua questa sottolineatura, ma ritengo che non lo sia nel dibattito culturale che si è sviluppato e si sta sviluppando soprattutto in questi ultimi anni sulle prerogative dei membri del Parlamento. Per chiedere il rispetto, che doverosamente bisogna chiedere, all'autorevolezza e libertà del Parlamento bisogna riuscire sempre a collocare questo tipo di discussione nella dialettica tra i poteri dello Stato e, se questa è la dialettica, rafforza anche l'autonomia degli altri poteri con cui andiamo a confrontarci in questa cornice istituzionale.

che il potere politico si collocasse non come potere in quanto tale, ma in questo tipo di dialettica. Oggi penso che il dibattito sia molto attuale, essendo anche mutato un quadro nazionale e internazionale delle forze in campo e con una grande possibilità di influenza e di determinazione della vita pubblica e privata dei cittadini. Signor Presidente, a nome del Gruppo Lega, preannuncio il voto favorevole alla Costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale.

Con riferimento alla fattispecie in esame, si è ritenuto all'unanimità che ricorressero tutte le condizioni indicate anche dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale per la configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità. Voglio ricordare in particolare che il suddetto tribunale ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica la valutazione della condotta addebitabile al senatore Esposito, in quanto estranea alla previsione di cui all'articolo 68 della Costituzione, richiedendo altresì l'annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato il 9 gennaio del 2019. Il principio della separazione dei poteri costituisce un postulato fondamentale di uno Stato democratico e presuppone, fin dai tempi dell'Illuminismo, una reciproca autonomia dei vari poteri: di quello legislativo, del quale interprete esclusivo è il Parlamento, di quello esecutivo ed infine di quello giudiziario. Tale prospettiva di fondo permea il sistema delle immunità, che svolgono proprio la funzione di prevenire o impedire intrusioni o sconfinamenti indebiti da parte dell'Autorità giudiziaria nelle prerogative del Parlamento. La Giunta, operando nel solco tracciato dalla stessa Corte costituzionale, ha confinato il sindacato del Senato ai soli profili di manifesta implausibilità ed altresì ai casi in cui tali profili emergano *per acta* senza necessità di accertamenti. Riportando quindi le parole dell'articolo 68 della Costituzione «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni», ritengo - come già anticipato anche a nome del Gruppo Lega - che è sicuramente configurabile la prerogativa dell'insindacabilità che il Senato dovrà difendere nel conflitto di attribuzione in questione. Prospetto pertanto la necessità che il Senato si costituisca in giudizio per far valere le proprie ragioni e le proprie prerogative.

Signor Presidente, colleghi e membri del Governo, oggi l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi in merito alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal tribunale ordinario di Torino, in relazione alla delibera con la quale in quest'Aula a gennaio è stata dichiarata l'insindacabilità per alcune dichiarazioni rese dal senatore, all'epoca dei fatti, Stefano Esposito, interpretando così l'articolo 68, primo comma, della Costituzione. L'azione oggetto della delibera furono le dichiarazioni pronunciate durante un'intervista radiofonica rilasciata nel gennaio del 2014 sugli scontri della TAV Torino-Lione. Nella predetta intervista Esposito, facendo riferimento ad un episodio intimidatorio di cui è stato vittima, indicò come potenziale mandante morale il dottor Livio Pepino, il quale lo denunciò per diffamazione aggravata a mezzo stampa. Ad un primo impatto si potrebbe ritenere che il Senato debba in ogni caso costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale per difendere le posizioni prese, a prescindere dal caso in esame, in maniera quindi automatica senza focalizzare l'attenzione sull'opportunità o meno di farlo. Noi del MoVimento 5 Stelle vogliamo invece spezzare questi automatismi dettati da vecchi equilibrismi politici e vogliamo invece analizzare il caso in maniera oggettiva ed approfondita per valutare le vere ragioni e l'opportunità di tale costituzione in giudizio, perché siamo convinti che dietro gli automatismi si possano nascondere scorciatoie e si possano accampare scuse per giustificare privilegi privilegi per la classe politica, a svantaggio dei semplici cittadini e, quindi, a svantaggio di giustizia e verità. Intanto mi permetto di ricordare a quest'Assemblea che la Corte costituzionale perimetra l'applicazione dell'esimente (quindi dell'immunità *ex* articolo 68) entro entro un confine ben definito che è il nesso funzionale. Il nesso funzionale consiste nel collegare le dichiarazioni e l'attività politica e parlamentare fatte in Senato con l'attività politica svolta al di fuori della sede deputata al dibattito. Per questo motivo le dichiarazioni *intra* ed *extramoenia* devono essere vicine nel tempo ed assimilabili nel contenuto. Traducendo il concetto in altre parole, il parlamentare non può avvalersi dell'immunità riconosciuta dalla Carta costituzionale per finalità diverse da quelle che dipendono dalla sua funzione; non può beneficiarne quindi per nascondere attacchi personali verso avversari politici o semplicemente verso chi ha opinioni diverse dalle proprie. Le dichiarazioni devono essere quindi vicine nel tempo. Lo erano? No, erano dell'anno precedente, più di sei mesi prima dell'atto avvenuto. Soprattutto, le dichiarazioni devono essere assimilabili A noi non sembra così vero che i discorsi fatti in Aula contrari alla Torino-Lione abbiano una sostanziale corrispondenza con l'accusa fatta all'ex magistrato di essere il mandante morale dell'attentato solo per il fatto di aver scritto un libro che sosteneva la tesi opposta a quella dell'allora senatore Esposito. In questo caso, è stata rivolta l'accusa di essere il mandante morale del posizionamento di bottiglie molotov davanti alla porta del senatore ad una persona che non era neppure un manifestante

di essere il mandante di un grave atto come quello di mettere in pericolo la vita umana con un'esplosione. Questa accusa specifica appare pertanto solo artificiosamente assimilabile nel contenuto all'attività parlamentare del senatore, come prevede l'articolo 68 della Costituzione. A questo punto, quindi, è necessario ragionare se riteniamo che sia opportuno che il Senato si debba costituire in giudizio davanti alla Corte costituzionale, che non vuol dire essere semplicemente presenti, ma vuol dire difendere la deliberazione presa, argomentare, sostenere la correttezza della concessione dell'insindacabilità, della concessione dell'immunità, insistendo per sottrarre al giudice la possibilità di un qualsivoglia giudizio sulle azioni commesse dal senatore Esposito, ripercorrendo l'approfondita valutazione che già facemmo mesi addietro. A gennaio, su queste basi, ravvisammo l'opportunità di non concedere l'immunità. Infatti l'Assemblea non si espresse all'unanimità per concederla, ma vi furono numerosi contrari, mi sembra di ricordare che furono 81. Di quei contrari, la quasi totalità (75) furono appunto del MoVimento 5 Stelle, ma anche ora restiamo fermi e continuiamo a non ravvisare, ora come allora, la sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni fatte in radio e quelle fatte in quest'Aula. Anche la recente giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 59 del 2018, ha stabilito che il tenore stesso delle frasi pronunciate dal parlamentare sia di per sé sufficiente ad escludere l'applicazione dell'insindacabilità dell'articolo 68, come non lo possono essere gli insulti e le diffamazioni solo perché in qualche modo collegati alle battaglie politiche di cui si fanno portatori i parlamentari. Lasciamo che la Corte costituzionale esamini gli atti, i resoconti di Giunta e la delibera del Senato, cosa che può fare già in assenza della parte resistente, avendo già tutti gli strumenti per valutare l'interpretazione della Costituzione Non insistiamo nello stiracchiare l'articolo 68 della Costituzione per trasformarlo in uno scudo di privilegi: quando si fa il parlamentare, si fa il parlamentare, ma fuori da questa funzione siamo tutti cittadini e siamo tutti uguali davanti alla legge. In conclusione, pertanto, colleghi, in merito alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica sul conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal tribunale ordinario di Torino, dichiaro il voto contrario del MoVimento 5 Stelle. Signor Presidente, non intendevo intervenire, ma diciamo che sono stato tirato per i capelli da un altro intervento.

è stata già abbondantemente esaminata prima in Giunta e poi nell'Aula del Senato. Mi pare davvero scorretto, quindi, richiamare l'attività del senatore Esposito che - lo voglio ricordare, perché nella scorsa legislatura io c'ero mille volte è intervenuto su quei temi in Aula e a causa dei suoi interventi è stato minacciato e vive tuttora sotto scorta per le minacce ricevute per sé e per i suoi bambini. Quindi richiamare qui l'attività del senatore Esposito mi pare davvero scorretto. Qui stiamo parlando di difendere le prerogative del Senato, che ha assunto una decisione che deve essere essere difesa nelle sedi competenti, rispettando i ruoli. *(Applausi)*. Finché - vivaddio - abbiamo un sistema democratico in Italia, anche davanti alla Corte costituzionale le parti che si presentano hanno diritto alla difesa; da una parte ci sarà chi ha impugnato, con i propri difensori, e dall'altra parte ci sarà il Senato, che giustamente si deve costituire per difendere le decisioni che erano state assunte. Quindi nessuna difesa delle prerogative; l'articolo 68 è un'altra cosa rispetto a ciò di cui stiamo parlando. Ne abbiamo già discusso e ne abbiamo già parlato; mi sembra che la questione si debba esaurire così. Annuncio pertanto il voto favorevole alla proposta di nomina di un avvocato davanti alla Corte costituzionale.

alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Torino, VI sezione penale. *(Segue la votazione)*.

Allegato B)*. La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, a uno o più avvocati del libero foro.

Signor Presidente, colleghi, intervengo per illustrare la relazione sull'emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti, approvata all'unanimità dalla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti lo scorso 8 luglio. Uno degli aspetti collaterali dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che è apparso da subito rilevante è stato quello relativo all'impatto che la pandemia avrebbe avuto sui rifiuti, sia in relazione alle conseguenze dell'azione di contenimento e contrasto della pandemia stessa che relativamente alle implicazioni che l'incremento massiccio nell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e dei diversi strumenti volti a fronteggiare e convivere con il coronavirus potevano comportare. Aspetti che si legano alla gestione dei rifiuti domestici ospedalieri e prodotti sui luoghi di lavoro. Si tratta di elementi che sono apparsi da subito rilevanti e in relazione ai quali i diversi soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti, in particolare le Regioni, hanno posto in essere una serie di azioni. A fronte di questa situazione, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlati ha ritenuto necessario un intervento tempestivo, al fine di approfondire quanto accaduto nei mesi di più acuta emergenza e di offrire al Parlamento, ai decisori pubblici e nei vari livelli di governo, al mondo produttivo e ai cittadini, un quadro di ciò che si è verificato e alcuni elementi utili in prospettiva futura nella gestione dei rifiuti cosiddetti Covid e non solo. Per quanto concerne il metodo di lavoro, oltre alla tempestività, l'altro elemento cardine che ha ispirato il modo di procedere della Commissione è stato quello della massima apertura all'ascolto e al recepimento delle indicazioni pervenute dagli interlocutori, identificati tra soggetti pubblici e privati con competenze nell'ambito del ciclo dei rifiuti, dal Ministero dell'ambiente a ISPRA, dall'Istituto superiore di sanità al Ministero della salute, dai rappresentanti del mondo associativo delle imprese di settore alla procura generale presso la Corte di cassazione. riguardo ai contenuti della relazione, dopo un inquadramento del contesto normativo generale dell'emergenza, il documento si concentra naturalmente sugli interventi in materia di rifiuti, un aspetto sul quale, al di là degli elementi di merito riportati in modo puntuale nella relazione, mi pare utile evidenziare in un'ottica propositiva che, dal punto di vista del metodo, è emerso l'utilizzo di fonti eterogenee, non sempre di natura normativa, nonché modalità e una dialettica di intervento tra Stato e Regioni rispetto alle quali potrebbero essere utili, in futuro, un maggior coordinamento e una minore propensione all'apertura rispetto a norme derogatorie. Passando agli effetti dell'emergenza epidemiologica sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti ricostruiti nella relazione, l'emergenza nella sua fase più acuta ha comportato una diminuzione della produzione dei rifiuti in generale, una diminuzione che però non ha alleggerito i *deficit* strutturali del sistema impiantistico nazionale che, anzi, hanno visto acuirsi gli effetti della carenza di possibili destinazioni per specifiche tipologie di rifiuti attualmente non gestite sul territorio nazionale per l'assenza di una specifica dotazione impiantistica ovvero di una filiera economica del trattamento della materia correttamente costruita. È poi importante sottolineare che, pur non avendo ovviamente alleviato i citati *deficit* strutturali, l'emergenza non ha prodotto interruzioni o alterazioni significative nella gestione dei rifiuti e le imprese e i lavoratori del settore, nonostante alcune fasi di difficoltà determinate da necessità di approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale, hanno concorso positivamente a interventi organizzativi tali da consentire il mantenimento di livelli adeguati di servizio. Gli effetti sulla produzione dei rifiuti e sulla loro gestione hanno dunque riguardato, in primo luogo, l'uso di materiali indotti dalla necessità di contenimento del contagio, suscettibili di produrre, sia un aumento della produzione dei rifiuti derivanti da materiali quali prodotti usa e getta nel commercio, nella ristorazione, nel confezionamento dei prodotti alimentari, sia fenomeni di abbandono diffuso, in particolare di mascherine facciali e guanti. A partire da questi elementi, che qui ho solo tratteggiato e rispetto ai quali rimando alla lettura del testo integrale della relazione, mi pare irrilevante sottolineare che, come in altri settori, per i rifiuti l'emergenza Covid ha rappresentato una sorta di lente di ingrandimento di dinamiche e aspetti strutturalmente presenti prima dell'emergenza e dei quali sarà necessario tener conto in prospettiva per interventi puntuali da parte di diversi soggetti competenti. Come evidenziato, infatti, quello che è emerso dall'inchiesta in termini di utilizzo di fonti eterogenee non sempre di natura normativa, dialettica a livello di intervento tra Stato e Regioni, caratteristiche e ahimè carenze, almeno sotto alcuni aspetti, dell'impiantistica e delle strategie nazionali della gestione dei rifiuti, non è evidentemente qualcosa di nuovo, ma qualcosa che, come anche nel caso del rischio di possibili fenomeni illeciti legati al ciclo dei rifiuti, l'emergenza ha reso e rende più evidente. Rimandando ancora una volta alla lettura del testo integrale, vorrei richiamarne alcuni aspetti di prospettiva, potremmo dire indicazioni di *policy*, evidenziati nella relazione. Innanzitutto, l'opportunità di considerare l'impatto economico dell'emergenza sulle tariffe e sugli introiti delle imprese e degli enti pubblici, con particolare riguardo alla sospensione della riscossione della Tari. In secondo luogo, la necessità di dedicare attenzione al mantenimento del rispetto dei principi nazionali ed europei in materia di economia circolare e degli obiettivi in questo campo, valutando con attenzione gli scenari attesi, anche in relazione a mutate abitudini di consumo e di organizzazione del lavoro e della produzione. Una necessità cui si è affiancata quella di affrontare il tema dell'*end of waste* in modo sistematico, rapido, con uno sguardo al futuro. Rilevante è poi l'esigenza di prestare un'attenzione particolare alla raccolta e al trattamento dei rifiuti ospedalieri, basati su incenerimento e sterilizzazione, che possono evolvere se le valutazioni tecnico-scientifiche sulla chiusura effettiva del ciclo saranno affiancate da adeguati interventi normativi che accompagnino verso soluzioni a minor impatto ambientale complessivo. Non meno rilevante è la necessità di promuovere l'esame scientificamente fondato e assistito dell'attività dei soggetti pubblici con competenze tecniche e scientifiche (Istituto superiore di sanità, ISPRA, luogo) dei temi della presenza di virus o materiale generico di virus nelle acque reflue e del rapporto tra emergenza epidemiologica e inquinamento atmosferico. Si tratta di due aspetti che sono stati approfonditi solo in maniera limitata nell'ambito della relazione, ma che certamente hanno significativi tratti di interesse sia per la Commissione sia, più in generale, per i soggetti che si occupano di ambiente e salute. Non possiamo poi dimenticare, come già più volte sottolineato, che le scelte di trattamento dei rifiuti e di chiusura del ciclo dei rifiuti, in relazione alla specificità dell'emergenza e del futuro atteso, dovranno considerare le criticità di segmenti del sistema impiantistico nazionale e la necessità di costruzione di una filiera economica nel trattamento in materia. Inoltre, l'adeguatezza della produzione normativa andrà misurata sulla capacità di integrazione tecnicamente e giuridicamente elevata tra norme statali primarie, norme statali secondarie, normativa regionale, tenendo conto dell'esperienza dell'emergenza epidemiologica e degli scenari futuri attesi, anche sulla base di un monitoraggio, affidato agli enti istituzionali, dell'evoluzione delle situazioni e della loro percezione diffusa. In questo senso, le norme derogatorie statali e le ordinanze derogatorie regionali dovranno essere superate. Ancora, l'emergenza epidemiologica ha amplificato la diffusa richiesta di semplificazione anche in materia di regolazione ambientale. L'accoglimento d'istanza in tal senso che dovesse riguardare i procedimenti amministrativi dovrà essere ponderata e compensata da un'adeguata pianificazione di controllo, che dovrà essere coordinata tra le agenzie di controllo ambientale e di controllo sanitario, polizia giudiziaria, ordinaria e specializzata, per non gravare su imprese e cittadini con controlli su controlli, bensì razionalizzando l'intervento pubblico. Non da ultimo, è bene sottolineare che la reazione a fatti illeciti e a possibili fenomeni illeciti dovrà avvenire sulla base del più ampio scambio di informazioni e di strumenti di coordinamento tra le autorità giudiziarie, nonché tra queste ultime e polizie giudiziarie ed enti di controllo. Infine, è importante richiamare il bisogno di un'opera di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui diversi aspetti che riguardano i rifiuti i rifiuti cosiddetti Covid e i rifiuti in generale, con l'obiettivo di ricondurre a razionalità l'uso dei presidi individuali e dei materiali usa e getta nonché la raccolta e il conseguente trattamento dei materiali dismessi. In questo modo si potrà costruire dal basso una strategia di sostenibilità che possa permetterci di guardare con maggiore speranza al futuro in termini ambientali ed economici: due elementi che o sono declinati insieme o semplicemente non sono.

Signor Presidente, come riferito dal relatore, dopo mesi di intenso lavoro, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha concluso - l'8 luglio 2020 - con l'approvazione della relazione sull'emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti. A nostro avviso si tratta di un lavoro importante, sul quale vogliamo esprimere un apprezzamento per il metodo che è stato seguito e per le modalità con le quali si sono svolti i lavori. Voglio ringraziare i relatori, i colleghi, gli Uffici e i consulenti della Commissione bicamerale, che hanno coadiuvato l'attività. Naturalmente l'auspicio per il Governo e per tutti gli enti è che facciano buon uso di questo studio e di questa attività di analisi che, a nostro avviso, ha chiarito molti aspetti di questo periodo particolarmente complicato e ovviamente inedito per Dopo un ampio ciclo di audizioni che ha visto la partecipazione del Ministero dell'ambiente, dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità, del Ministero della salute e dei rappresentanti del mondo associativo delle imprese del settore, oltre alla procura generale presso la Corte di cassazione, è stato tracciato un quadro completo dell'impatto che l'emergenza Covid ha avuto nel campo della gestione del ciclo dei rifiuti, facendo emergere una chiara esigenza di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché l'esigenza di sicurezza per i lavoratori del settore e l'esigenza di implementazione dell'impiantistica, oltre ad una necessità di elevata attenzione a possibili fenomeni criminali che si muovono a margine di un'economia legale naturalmente fortemente in crisi per gli accadimenti connessi all'emergenza epidemiologica. un lavoro che noi riteniamo soddisfacente e che rappresenta un importante contributo che il Parlamento offre all'azione di Governo perché analizza in tutti i suoi aspetti l'impatto che ha avuto l'emergenza La relazione, a nostro giudizio, è approfondita su moltissime e delicate questioni che vanno dalla ricostruzione del quadro normativo in cui ci si è mossi fino agli interventi in materia di rifiuti agli effetti che si sono generati sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti, senza tralasciare le questioni riguardanti l'uso dei presidi individuali di protezione e i rifiuti sanitari. Molta attenzione è stata focalizzata anche sull'impatto ambientale di forme di sanificazione diffusa, sul trattamento delle acque reflue e il possibile rapporto tra inquinamento atmosferico e contagio. attenzione è stata dedicata alla cura della cultura e della legalità, per tenere alta la guardia verso una criminalità che da sempre cerca di insinuarsi nel ciclo dei rifiuti, soprattutto nei momenti di emergenza che possano interessarlo. Naturalmente ci attendiamo che il Governo faccia buon uso di questo prezioso lavoro, facendo seguire all'analisi la terapia. Fratelli d'Italia ha sottoscritto e voterà pertanto a favore della risoluzione unitaria che è stata presentata. In particolare vogliamo sottolineare due impegni che vengono sottoposti al Governo: il primo riguarda la fine del rifiuto. da molto tempo stiamo sollecitando il Ministero affinché questa realtà trovi un suo compimento. Lo riteniamo assolutamente fondamentale. Come convenuto con il collega Zaffini che avrebbe dovuto tenere il suo intervento in discussione generale, riteniamo molto importante anche affrontare le criticità dei segmenti del sistema impiantistico nazionale per il trattamento dei rifiuti e di chiusura del ciclo dei rifiuti, in relazione alle specificità dell'emergenza e del futuro atteso e alla necessità di costruire una filiera economica del trattamento della materia, oltre poi alla chiusura della risoluzione che riguarda il sistema dei dei controlli. Riteniamo infatti che ci sia un'esigenza vera e concreta di un coordinamento tra le diverse agenzie e i diversi enti, per fare in modo che non ci siano controlli su controlli, che finiscono soltanto per vessare gli imprenditori seri di questo settore. L'esperienza

ribadendo al Governo la necessità di un impegno preciso e forte per governare il ciclo di rifiuti, perché, in questi anni, di risultati e di avanzamenti ne abbiamo visti ben pochi.

la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati relativa alla "emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti", approvata all'unanimità una lente d'ingrandimento, che consente di verificare una serie di aspetti legati al ciclo dei rifiuti, ai suoi problemi e anche alle connessioni, che purtroppo

sia esaustiva e che metta in luce anche alcune criticità, che non sono limitate alla gestione dei rifiuti legati alla pandemia, ma che riguardano problemi, che dovrebbero essere affrontati in senso generale nella gestione dei rifiuti. Restando alla relazione specifica sull'emergenza epidemiologica e il ciclo dei rifiuti, riteniamo che il lavoro della Commissione, che ha potuto beneficiare di numerose audizioni, dalle agenzie, alle associazioni, alle imprese che si occupano di queste attività, finanche alla procura generale

dovrà intervenire. Con la risoluzione presentata, si chiede appunto di poter operare in questa direzione. C'è un tema legato ad un adeguato livello di gestione dei rifiuti, in senso complessivo, ma soprattutto c'è una questione legata al rapporto e alla dialettica tra lo Stato e le Regioni: se non si va ad operare in maniera adeguata ed efficiente in questo rapporto, rischiamo di non poter incidere in maniera positiva e significativa sul livello di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali stessi. C'è un tema legato all'impiantistica, con alcune carenze che sono state evidenziate nell'indagine della Commissione, insieme al riflesso e all'impatto economico che hanno sulle tariffe. C'è poi un tema specifico, che riteniamo essere tra i più rilevanti e importanti, che è quello della ricerca di soluzioni a minor impatto ambientale. Oggi i rifiuti di carattere sanitario vengono tutti inceneriti, con le conseguenze che ben conosciamo. Sappiamo che sono in corso ricerche e studi, per poter gestire in maniera più

delle ricerche e degli investimenti in tecnologia, per promuovere procedure e la creazione di impianti che, come dicevo, siano maggiormente sostenibili da un punto di vista ambientale. Su questo consentitemi di dire che, anche in una recente discussione che è stata fatta in quest'Aula sul tema del glifosato, non sempre abbiamo avuto la capacità di rimetterci al ruolo della scienza in maniera corretta. Nella relazione in esame e nel lavoro fatto da questa Commissione è esplicitata in maniera chiara l'importanza di promuovere l'esame scientificamente fondato e assistito per poter prendere delle decisioni; nell'altra occasione quest'Assemblea si è divisa su posizioni molto diverse,

proceda nella direzione indicata dalla Commissione, ma che anche quest'Assemblea sappia sempre più farsi carico delle proprie responsabilità e delle azioni da intraprendere facendo riferimento alla verità che la scienza ci può fornire. In questo caso attenderemo che le ricerche in corso e gli investimenti che si stanno compiendo possano fornire al Governo tutti gli utili elementi per poter andare nella direzione di un diverso trattamento dei rifiuti di carattere sanitario.

di controlli su controlli, facendo sentire tutto il peso di queste procedure. Ancora una volta, dunque, emerge in tutta evidenza l'esigenza per il nostro Paese di semplificare, che non vuol dire voltarsi da un'altra parte e non guardare cosa accade, atteso che i controlli necessari, anche in questo ambito così delicato, possono essere fatti semplificando le procedure e non costruendo orpelli burocratici che poi giustificano soltanto il fatto che qualcuno debba operare e far girare delle carte. I controlli sono necessari, ma, come insegnano anche le esperienze di altri Paesi, possono essere svolti e compiuti in maniera

principali, quella di studio e analisi dei fenomeni che si vengono a determinare, sottoporre ai legislatori, al Parlamento o anche al Governo, le problematiche con dei suggerimenti di soluzioni. Questa è una delle sue prerogative più importanti e l'ha subito messa in atto

perché emergesse un quadro il più chiaro possibile della situazione. Chiaramente il Covid-19 è stato per tutti i livelli un fatto nuovo e inaspettato, difficile da gestire con cognizione, perché non si sapeva cosa fosse, quindi possiamo dire che abbiamo dovuto affrontare almeno tre fasi: nella prima era necessario ridurre l'impatto del virus, salvare immediatamente le vite a qualunque costo;

futuro. Nella prima fase si sono commessi anche molti errori di valutazione e gestione, come per esempio quello di dare la delega alle Regioni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti con le ordinanze regionali: questo ha creato sovrapposizioni, confusioni e mancanza di omogeneità, che riteniamo uno dei punti a cui si deve porre rimedio. Si è creduto che si sarebbero prodotti più rifiuti e infatti un articolo del decreto prevedeva l'aumento della potenza dell'impiantistica, che poi fortunatamente è stato cancellato nel decreto rilancio alla Camera, perché non sono stati prodotti più rifiuti, anche perché nel bilancio complessivo il *lockdown* ha creato un decremento della loro produzione.

l'attitudine dei cittadini ad avere o meno una corretta gestione dei rifiuti. Adesso però ci troviamo nella fase in cui è necessario ridurre l'impatto della produzione dei rifiuti e il conseguente carico ambientale. grazie a tutti dopo un primo momento in cui hanno dovuto riorganizzare la loro attività, sono stati all'altezza dei loro compiti. Ci troviamo però alle prese con nuovi prodotti,

dalle esalazioni che vengono dal parlato, dallo starnuto e via di seguito. Il ministro Costa aveva auspicato

che rientrano anche nella semplice disposizione normativa. Questo quindi è un auspicio che cogliamo, su suggerimento del Ministro, per migliorare e dare la possibilità in futuro di produrre

ossia se la mascherina viene usata da un soggetto sicuramente contagiato è un

perché è stato dimostrato che il cibo non è trasmettitore del virus e quindi tutto il monouso, utilizzato anche nell'impacchettamento dei generi alimentari, è assolutamente inutile. Allo stesso modo, i disinfettanti possono possono essere gli aggravanti dell'inquinamento delle acque reflue laddove non sono così necessari, come invece creduto normalmente da parte della popolazione; basta un lavaggio frequente. frequente. Ci troviamo in una situazione in cui potremmo dire che il gatto si morde la coda, perché stiamo affrontando un'emergenza sanitaria causata da un virus che è favorito - come è stato accertato dall'inquinamento e dai cambiamenti climatici e, con la produzione di monouso e plastiche anche laddove non necessaria,

una correlazione causa-effetto. È stato accertato che, laddove c'è maggiore concentrazione di PM2,5 e PM10, c'è anche una predisposizione, probabilmente perché gli individui hanno già un'infezione polmonare che peggiora la loro ricettività al virus.

di uso sanitario c'è necessità di un miliardo di mascherine al mese. La plastica contribuisce in maniera drammatica al cambiamento climatico e disperde nell'ambiente gas serra. Da uno studio del CIEL,

In due mesi di attività molto serrata abbiamo avuto modo di incontrare molti mondi: esperti, istituzioni, rappresentanti di associazioni e categorie

In particolare, è stato molto utile il rapporto stretto e organico che abbiamo mantenuto costantemente con l'Istituto superiore di sanità, piuttosto che con l'ISPRA. È stato dunque un grande lavoro comune,

È già stato sottolineato come durante la pandemia vi sia stato certamente un aumento, di circa 200.000 tonnellate, di rifiuti legati rifiuti legati ai dispositivi di protezione individuale, in particolare di mascherine e di guanti. A fronte di questo, il sistema ha retto; il sistema nazionale ha retto non certo perché vi sia un piano organico e di distribuzione capillare per affrontare in maniera adeguata la gestione e la chiusura del ciclo dei rifiuti nel nostro Paese (anzi, tutt'altro), ma semplicemente perché l'aumento di 200.000 tonnellate dei dispositivi di protezione individuale è stato esattamente pari alla diminuzione di rifiuti organici e non organici (quindi di rifiuti urbani) nel nostro Paese.

Signor Presidente, ho solamente alcune sottolineature in questo quadro assolutamente importante dal punto di vista della collaborazione e della collegialità politica, con riferimento a questa risoluzione che vede la firma non solo del Partito Democratico e del sottoscritto, ma di tutti. Alcune raccomandazioni al Governo: incidere in maniera significativa e ancor di più sull'economia circolare; noi lo stiamo facendo. Alcune settimane fa in Commissione ambiente abbiamo terminato un lavoro, durato tre mesi,

Nel 2019 la legge di delegazione europea ha stabilito il quadro della norma generale e, all'interno di questo, lo schema di decreto legislativo predisposto dal Ministero dell'ambiente è stato elaborato dalla Commissione competente, caso con soddisfazione. Tre di questi quattro provvedimenti, che modificano in maniera strutturale il sistema della gestione dei rifiuti, dei veicoli usati, delle discariche e una parte consistente del testo unico sull'ambiente, sono stati votati fondamentalmente senza voti contrari, nemmeno dell'opposizione. Questo per dire che il Senato ha lavorato in questa direzione e dunque si è fatto trovare pronto anche a quanto emerso nell'emergenza da Covid-19.

La presente risoluzione prende in considerazione la tecnologia e l'organizzazione come fattori positivi per la gestione del ciclo dei rifiuti, in emergenza e fuori dall'emergenza. è stato, poi, un approfondimento molto interessante sulla presenza di virus o di materiale genetico del virus nelle acque reflue. È un indicatore di grande evidenza scientifica e di grandi conseguenze, che naturalmente non sfuggono a nessuno di noi, dal punto di vista delle ricadute per la saluta pubblica. Vi è stato un approfondimento altrettanto importante anche nella relazione tra la crisi, la pandemia e l'inquinamento atmosferico. Ora, per sfrondare polemiche inutili e dubbi, diciamo subito due cose: la relazione stabilisce che è sufficientemente provato il rapporto tra inquinamento atmosferico elevato, pressione ambientale sulle popolazioni e suscettibilità maggiore a un'infezione batterica o virale, in particolare derivante da patologie croniche legate ad elevata concentrazione di particolato. È, dunque, scientificamente provata una correlazione tra l'inquinamento e la diffusione dei virus e, quindi, del Covid-19. È, invece, da approfondire il meccanismo attraverso il quale questa pandemia si può diffondere. È provata la sovrapposizione tra il massimo sviluppo della pandemia e le aree fortemente inquinate a livello mondiale,

che coinvolge numerose ARPA regionali in modo da approfondire la questione. Unitamente a queste, sulla relazione tra pandemia e ambiente non vi è dubbio alcuno, dal punto di vista fenomenologico, che vi sia una relazione diretta tra la deforestazione, lo *sprawl* urbano, il contatto tra uomo e animale e, dunque, la diffusione dei virus, perché è noto che il virus è stato portato da animali non domestici all'uomo. Questa vicinanza, che prima non esisteva, è dovuta in maniera evidente agli elementi di cui parlavo prima. Di conseguenza, non c'è dubbio alcuno,

che c'è una relazione diretta tra il cambiamento del clima, l'azione antropica e la diffusione dei batteri e del virus a livello mondiale.

il lavaggio delle mani. Da parte di quasi tutti è stato messo in evidenza che l'utilizzo di guanti deve essere riservato agli operatori dei settori e c'è anche una sottolineatura importante sul fatto che è inutile usare stoviglie usa e getta di plastica. Sono del tutto sufficienti una sana igienizzazione e un lavaggio. Un altro punto importante è stata l'individuazione la centratura del ragionamento sui rifiuti ospedalieri attualmente basati su incenerimento e sterilizzazione. Presidente, vi è, infine, la questione del sistema impiantistico. questa epidemia ha messo in evidenza che c'è una forte criticità e c'è bisogno di lavorare in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale perché il trattamento dei rifiuti ha bisogno di una sana politica industriale di impianti

dal primo giorno dell'avvio dello stato di emergenza a seguito della pandemia - periodo che personalmente ho vissuto a Bergamo nella mia città, nel cuore della mischia - la prima preoccupazione o, anzi, la paura vera e propria è stata quella che potesse fermarsi il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Per questo ho verificato in maniera sistematica le condizioni delle aziende preposte e del personale e degli operatori, veri e propri eroi un po' dimenticati, senza i quali però sarebbe potuta essere una tragedia nella tragedia. Neanche per un giorno si sono fermati, nonostante la carenza di presìdi, di mascherine e di protezioni a volte. Ogni giorno, affacciata al mio balcone, quel balcone da cui ho visto passare i camion con le bare dei miei concittadini, tra cui molti amici, mentre il Covid si era insinuato perfino in casa mia, ogni giorno ho gridato grazie e mandato un bacio a quegli uomini e quelle donne che, nel silenzio delle strade deserte, passavano a raccogliere i sacchi e il loro contenuto pericoloso senza paura e con altissimo senso del dovere. Scusate, ma ci tenevo, in apertura della dichiarazione di voto di Forza Italia, a rinnovare tutta la nostra riconoscenza per chi, invisibile ma indispensabile, ha consentito che le città e i paesi non si riempissero di rifiuti scatenando pandemia nella pandemia nel momento più terribile. Grazie, grazie e ancora grazie. Uno degli aspetti collaterali all'emergenza sanitaria Covid infatti, forse quella realmente più pericolosa, è stato quello relativo all'impatto che la pandemia avrebbe avuto sui rifiuti, sia in relazione alle conseguenze alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia stessa, che rispetto alle implicazioni che l'incremento massiccio dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, di mascherine e di guanti soprattutto, avrebbero potuto comportare. La gestione dei rifiuti ha avuto un'impennata di difficoltà, ma nessuno se ne è accorto accorto grazie all'organizzazione e alla fermezza con cui si è rimasti sul pezzo. Gestione dei rifiuti domestici, gestione dei rifiuti ospedalieri, gestione dei rifiuti prodotti sul posto di lavoro: per i territori maggiormente colpiti, come la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e l'Emilia Romagna è stato veramente un periodo incredibile, surreale e consentitemi di dedicare un pensiero ai negazionisti che, buon per loro, probabilmente non sono stati colpiti come sono state colpite le Regioni del Nord. Tornando alla le Regioni del Nord. Tornando alla gestione del ciclo dei rifiuti tutti i soggetti coinvolti in particolare le Regioni, le Provincie e i Comuni, hanno subito reagito ponendo in essere ogni azione necessaria a contenere la pandemia assicurando il miglior servizio possibile ai cittadini. Quello che oggi la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha prodotto è una relazione, a cui si affianca una risoluzione firmata da tutti i Gruppi Gruppi - ripeto tutti e sottolineo tutti i Gruppi politici rappresentanti del Paese in Parlamento - un insieme di proposte concrete, condivise, utili, necessarie che derivano dall'intervento tempestivo della Commissione stessa al fine di approfondire quanto accaduto nei mesi di emergenza più acuta per offrire al Parlamento, ai decisori pubblici ad ogni livello di governo, al mondo produttivo e ai cittadini tutti, un quadro di ciò che si è verificato e alcuni elementi utili su cui ragionare e, possibilmente, intervenire

oggi, memori di quanto è successo, tutto il sistema della gestione dei rifiuti va rivisto trasformando (anche per questo comparto) una emergenza tragica in un'opportunità per migliorare le attività in un settore, spesso non considerato quanto si dovrebbe, levando paletti ideologici e superando concezioni antistoriche e integraliste senza senso. La Commissione ha lavorato come dovrebbe lavorare ogni Dicastero del Governo e *in primis* il Presidente del Consiglio: in un clima di massima apertura

rifiuti, dal Ministero dell'ambiente a ISPRA, dall'Istituto superiore di sanità al Ministero della salute, dai rappresentanti del mondo associativo delle imprese di settore alla procura generale presso la Corte di cassazione. perché questo è il lavoro serio e competente del Parlamento. Altro che inutili *task force*! E il nostro auspicio è che una risoluzione unitaria, che sarà votata all'unanimità, non faccia la fine di altre relazioni. Ciò che è stato evidenziato è quello che noi sistematicamente sosteniamo: dal punto di vista del metodo, occorrerà in futuro un maggior coordinamento tra Stato e Regioni, ricorrendo sempre meno all'apertura a norme derogatorie derivanti da fonti eterogenee non sempre di natura normativa. Per quanto riguarda l'effetto, l'emergenza ha comportato una diminuzione della produzione dei rifiuti in generale, una diminuzione che però non ha alleggerito i *deficit* strutturali del sistema impiantistico nazionale che, anzi, al contrario, hanno visto acuirsi gli effetti della carenza di possibili destinazioni per specifiche tipologie di rifiuti attualmente non gestite sul territorio nazionale per l'assenza di una specifica dotazione impiantistica, ovvero una filiera economica di trattamento della materia correttamente costruita; in parole povere: la carenza di impianti e la disomogeneità della loro presenza sui vari territori che ancora oggi fa sì che ci siano due Italie anche da questo punto di vista. Inconcepibile. A maggior ragione sottolineo ancora che, nonostante la carenza di impianti e la disomogeneità della loro presenza sui vari territori, l'emergenza non ha prodotto interruzioni o alterazioni significative nella gestione dei rifiuti grazie a Dio e grazie all'organizzazione delle imprese e dei lavoratori del settore - malgrado la difficoltà determinate dalla necessità di approvvigionarsi dei dispositivi di protezione individuale e malgrado la confusione prodotta dal commissario Arcuri, tutto è andato bene e i livelli adeguati di servizio sono stati mantenuti. Da evidenziare comunque il fenomeno di abbandono diffuso di mascherine e guanti che andrà perseguito in ogni modo possibile. Resta il fatto che l'emergenza ha fatto da "lente di ingrandimento" su quanto funziona e quanto non funziona, e questo a prescindere

di esami scientificamente fondati da ISS e ISPRA in primis, che grazie alle loro competenze tecniche, dovrebbero analizzare la presenza di virus o materiale genetico di virus nelle acque reflue; così come stabilire scientificamente il rapporto tra epidemia e inquinamento atmosferico, che potrebbe essere una delle spiegazioni della maggiore incidenza del virus proprio nella Pianura Niente di nuovo sotto il sole quindi, ma temi che vanno affrontati ora, subito, se vogliamo veramente essere efficaci rispetto al depotenziamento del rischio di possibili fenomeni illeciti legati al ciclo dei rifiuti che semmai l'emergenza ha reso ancora più evidenti. Vogliamo semplificare una volta per tutte - e ve lo chiederemo ancora all'interno del prossimo decreto semplificazione - ogni azione volta a realizzare davvero quel *green deal* che l'Europa ci chiede, ma che noi vogliamo profondamente per il bene e il benessere dei cittadini e dell'ambiente. Un Paese responsabile e moderno deve poter disporre di un sistema di gestione dei rifiuti adeguato ed evoluto sul piano industriale, e quindi della necessaria impiantistica per rispondere alle esigenze che emergono da una pianificazione del settore. Un sistema moderno è indispensabile per una adeguata gestione ambientale,

richiamo ad una forte attenzione al sistema dell'*end of waste* e alla semplificazione. Noi produrremo ancora emendamenti che ci auguriamo verranno presi in considerazione e approvati, perché solo così ne usciremo. Nell'annunciare il voto favorevole di Forza Italia alla relazione e alla risoluzione, vi chiedo ancora un forte applauso per tutti gli operatori del settore dei rifiuti, senza il cui senso del dovere oggi ci troveremo in una situazione molto più difficile. Grazie davvero.

tutti i colleghi hanno anticipato che sulla proposta di risoluzione ci sarà un voto unanime, e non perché tutto vada bene, ma perché i problemi che abbiamo riscontrato sono così evidenti che hanno imposto a tutti di individuare e suggerire al Governo degli interventi che possano evitare che il nostro Paese possa trovarsi di nuovo - Dio non voglia - di fronte a un'emergenza in modo così inadeguato e inappropriato anche nel settore della gestione dei rifiuti. Il fatto che le cose non siano andate peggio e che il sistema abbia tenuto non significa che significa che non si sarebbe potuto agire meglio. I Presidenti di Camera e Senato avevano chiesto a ogni Commissione, nella fase più calda dell'emergenza, di continuare a lavorare e di interrogarsi, per quanto di competenza, sulle conseguenze e studiare le possibili azioni che si sarebbero potute intraprendere in Parlamento per venire incontro alle esigenze del Paese. Ebbene, come Commissione bicamerale sugli ecoreati non ci siamo sottratti.

- è stato detto per la sanità e per l'inquinamento - che il quadro di partenza condizioni poi tutto il resto. E qual è il quadro di partenza che occorre ribadire ancora una volta? Sentirete questo fino

anche la comunicazione che c'è stata non ha aiutato, e ciò è emerso dai resoconti stenografici delle audizioni anche della parte privata, oltre che di quella pubblica. Pensate che, nonostante le infinite conferenze stampa, le infinite dichiarazioni e gli infiniti esempi del Presidente del Consiglio, mai una volta sono stati ricordati gli operatori; mai una volta è stato fatto l'esempio della gestione del ciclo dei rifiuti come di un servizio essenziale per evitare che un eventuale blocco potesse comportare il determinarsi di un'emergenza nell'emergenza. Per settimane, in alcuni casi per mesi, nonostante più volte il Presidente del Consiglio ci abbia ricordato che il 31 gennaio sia stato approvato lo stato d'emergenza, ancora a marzo le associazioni di categoria chiedevano chiarimenti e risposte. Cosa è arrivato a distanza di settimane o addirittura di mesi? Sono arrivate delle linee guida. Di fronte a domande specifiche rivolte tanto al Ministro della salute che a quello dell'ambiente, balbettando ci è stato detto che effettivamente

c'è la risposta della Regione Lombardia che specifica l'inquadramento dell'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'emergenza - ma potrei prendere anche l'esempio delle altre diciannove Regioni o delle Province autonome prima che una risposta arrivasse in maniera definitiva, con l'indicazione ad esempio dei codici Ateco degli impianti quali attività indispensabili. Ci si poteva muovere sicuramente prima. È ottimo ottimo prendere atto, anche per l'emergenza attuale e per il futuro, al punto 2 della proposta di risoluzione che è stata elaborata e nella quale ci riconosciamo pienamente, dell'esigenza di contemperare

che non era stato ancora richiamato nei precedenti interventi. Ben venga anche che si richiami il Governo sulla necessità di dare risposte sull'*end of waste*, sul ciclo dei rifiuti e sull'impiantistica,

direttive europee che abbiamo recepito - mi riferisco in particolare all'Atto Senato 169, che recepiva le direttive nn. 851 e 852 relative agli imballaggi e alla produzione di rifiuti - non ci sia stato nessun voto contrario. Responsabilmente, infatti, abbiamo guardato a quello che c'era di buono, ma abbiamo anche segnalato quello che si sarebbe potuto fare e non si è fatto. Faccio un unico esempio: chiedere di avere delle risposte, ridurre la produzione di rifiuti, aumentare il riciclo e poi imporre - chiedo un minimo di attenzione, perché è un passaggio importante, e mi rivolgo anche al Governo, perché fa ancora in tempo a correggere lo schema di decreto di decreto legislativo - gli *standard* minimi solo per gli impianti che preparano il rifiuto al riciclo. Vogliamo dire una volta una volta per tutte che ogni impianto rifiuti deve avere degli *standard* minimi per evitare quelle truffe legalizzate che spesso succedono in varie parti d'Italia e che sono oggetto anche delle indagini della Commissione bicamerale d'inchiesta? Ci sono degli impianti all'interno dei quali i rifiuti girano per finta solo per giustificare che, essendo scarti

completare la rete impiantistica, che non è presente in tutto il territorio nazionale, ma serve che quegli impianti funzionino sul serio e non sulla carta. Anche questo significa ridurre gli spazi per la criminalità, per il malaffare, per chi vuole speculare sui rifiuti. Prendiamo anche atto positivamente del fatto che la relazione riconosca la necessità di provvedere a garantire una quantità sufficiente dei nostri impianti di lavorazione. È infatti vero

sono state quelle prodotte e quelle trattabili, non sarebbero bastate. Allora una buona volta diamo una risposta. Una cosa è certa: l'unica emergenza legata attualmente al Covid per questo settore - a parte quella democratica che purtroppo - è l'assenza di un piano di gestione delle emergenze. Noi speriamo che possa finalmente essere approvato affinché, alla prossima occasione in cui il nostro Paese si troverà in difficoltà, si possa rispondere in maniera tale che questa emergenza non sia dimenticata, ma costituisca il punto di partenza per gestire ancora meglio la prossima, che speriamo non ci sia o sia il più lontano possibile. Signor Presidente, colleghi, nei mesi scorsi la gestione del ciclo dei rifiuti si è collocata in un quadro generale di problemi determinati dall'emergenza epidemiologica, le cui caratteristiche sono tali da incidere su aspetti sanitari ed economici, ma anche sui costumi sociali e sulla capacità di risposta nel settore dei servizi essenziali, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti, dalla raccolta al trattamento. Va considerato, in ogni valutazione da compiere sugli eventi verificatisi a partire dal gennaio 2020, che la stessa comunità scientifica mondiale si è trovata di fronte a un'assoluta novità. Le conoscenze si sono consolidate solo nel corso del tempo attraverso il dibattito pubblico della comunità scientifica e con la ricerca ancora in corso. La Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha ritenuto di interloquire in tempi rapidi con soggetti pubblici e privati e di concludere con la presente relazione un approfondimento sul tema "Emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti", al fine di fornire al Parlamento, agli organi di governo statali e regionali, al mondo produttivo e ai cittadini un quadro di quanto successo, nonché valutazioni e raccomandazioni orientate al futuro. Il contesto normativo generale di gestione dell'emergenza si presenta come di particolare complessità con fonti di livello diverso, statali, regionali e relative agli enti locali. In questo ambito ampio, le fonti in materia di ciclo dei rifiuti e di ambiente sono limitate, riducendosi a livello primario agli articoli 113 e 113*-bis* - peraltro quest'ultimo successivamente abrogato da un emendamento presentato dal MoVimento 5 Stelle - del decreto-legge n. 18 del 2020, che peraltro introducono norme derogatorie di portata generale, nonché all'articolo 30*-bis* del decreto-legge n. 26 del 2020, che interviene incidentalmente sul regime dei rifiuti sanitari. Non riguarda in sé il ciclo dei rifiuti, ma apre una prospettiva più ampia nel campo della tutela ambientale, l'articolo 4*-bis* del decreto-legge n. 23 del 2020, che ha inserito i servizi ambientali e le attività di bonifica nella lista delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione criminale. Sulla gestione dei rifiuti sono state fornite indicazioni e soluzioni di tipo scientifico e tecnico in relazione alla raccolta e al trattamento dei rifiuti, sulla base di un'apprezzabile collaborazione tra l'Istituto superiore di sanità e il Sistema nazionale di protezione ambientale. Gli interventi sul ciclo dei rifiuti sono, invece, in buona parte derivati da ordinanze delle singole Regioni, di natura derogatoria rispetto a regole vigenti, a cui va associata una circolare del Ministero dell'ambiente che ha suggerito alle Regioni stesse l'uso di ordinanze, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente). L'emergenza sanitaria non ha aumentato in maniera decisiva la produzione di rifiuti in generale; anzi, come diceva il senatore Ferrazzi, l'ha diminuita a causa del minor consumo di beni durante la fase di blocco i provvedimenti assunti hanno dato risposta alla percezione di *deficit* strutturali del sistema impiantistico nazionale, che nella fase dell'emergenza hanno acuito gli effetti della carenza di possibili destinazioni per specifiche tipologie di rifiuti, attualmente non gestite sul territorio nazionale per l'assenza di una specifica dotazione impiantistica ovvero di una filiera economica di trattamento della materia, correttamente costruita. La temporanea criticità derivante dalla chiusura di alcuni mercati esteri non segnala un'emergenza, bensì la circostanza che allo stato vi sono alcune esportazioni di rifiuti razionali in una logica di mercato globale e altre, invece, frutto della mancanza di impianti dedicati o conseguenti raccolta di rifiuto scadente: ciò rende necessario, in prospettiva, anche a breve e medio termine, creare le condizioni normative ed economiche per investimenti in innovazione ambientale compatibile. L'emergenza sanitaria non ha prodotto interruzioni e alterazioni significative nella gestione dei rifiuti: le imprese e i lavoratori del settore, nonostante alcune fasi di difficoltà determinate dalla necessità di approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale, hanno concorso a consentire il mantenimento di una risposta adeguata al servizio. Va apprezzato l'orientamento tendente a non proclamare alcuno stato di eccezione, mantenendo, invece, indicazioni coerenti con le norme vigenti per la classificazione dei rifiuti e riconducendo ad esso le esigenze della fase emergenziale anche in considerazione di quanto sinora noto scientificamente sulla limitata persistenza del virus sulle superfici. L'ISPRA ha costantemente informato e aggiornato in tal senso gli enti locali. L'emergenza epidemiologica ha generato effetti - ed è destinata a generarne - sulla produzione dei rifiuti, con conseguenze sulla loro gestione che riguardano sia la produzione generale sia quella derivante dall'uso di specifici prodotti destinati al contenimento del contagio. A questo proposito, i temi rilevanti riguardano l'uso di materiali indotti dalla necessità di contenimento del contagio stesso, suscettibili di produrre un aumento nella produzione di rifiuti e fenomeni di abbandono diffuso: faccio riferimento all'uso delle mascherine facciali e dei guanti, ma anche dei materiali "usa e getta" nel commercio, nella ristorazione e nel confezionamento dei prodotti alimentari. Come sottolineava la senatrice Nugnes, spesso e volentieri questi materiali "usa e getta" sono inutili ai fini del contenimento del contagio. Nell'ambito dell'emergenza epidemiologica, tra le azioni volte al contenimento è risultato ampiamente diffuso l'utilizzo di mascherine facciali di vario tipo e di guanti, anche nelle azioni quotidiane non direttamente collegate ad attività lavorative. Le disposizioni in materia sono state plurime, provenienti da fonti statali, regionali o locali con specifiche ordinanze che si sono evolute nel tempo ma, sottolineo, alcune volte anche contraddette tra di loro. Un secondo tema rilevante riguarda gli scenari della produzione di rifiuti determinata nelle fasi di nuova normalità, dopo l'emergenza epidemiologica, con particolare riguardo ai rifiuti solidi urbani e ai rifiuti sanitari. Vi sono poi questioni correlate di cui la Commissione d'inchiesta ha ritenuto di occuparsi: si tratta dell'impatto ambientale di forme di sanificazione diffusa, del trattamento delle acque reflue e del possibile rapporto tra inquinamento atmosferico e contagio. La Commissione ha acquisito dagli interlocutori dagli interlocutori individuati durante l'inchiesta, in particolare - per quanto riguarda i presupposti scientifici - dall'Istituto superiore di sanità, dal Ministero della salute e dall'ISPRA, le evidenze necessarie a fornire alcune raccomandazioni, sulla base di quanto finora noto, circa l'evoluzione del contagio, le valutazioni devono distinguere gli effetti legati alla prima fase dell'emergenza dagli effetti di medio periodo conseguenti al superamento dei picchi di contagio e di necessità di cura e legati al potenziale emergere di nuove Se in una prima fase dell'emergenza la priorità assoluta è stata quella di salvare vite, ridurre l'impatto del contagio ed evitare il collasso del sistema sanitario e dei sistemi sociali che una diffusione esponenziale dei contagi avrebbe prodotto, adesso si pone il tema di avviare la ricerca scientifica, l'elaborazione tecnologica e l'innovazione organizzativa delle imprese e della pubblica amministrazione verso soluzioni che portino alla riduzione dei rifiuti e, più in generale, ad investimenti sulla tutela dell'ambiente e sulla sostenibilità ambientale.

andrà considerato, altresì, l'impatto economico dell'emergenza sulle tariffe, con particolare riguardo alla sospensione della riscossione della Tari. Nella fase più acuta dell'emergenza epidemiologica, l'uso dei dispositivi individuali di protezione e di materiali usa e getta, come detto, hanno posto a confronto la percezione del rischio, l'ansia di ipotesi risolutive e, al contrario, la necessaria e lungimirante valutazione del saldo sanitario e ambientale complessivo delle azioni intraprese; su questo confronto, la Commissione ritiene, sulla base della trasmissione interumana del coronavirus, che la funzione delle mascherine facciali, come dispositivi destinati a proteggere le altre persone, può essere assolta da mascherine chirurgiche utilizzate in forma anche alternata o protratta, ovvero da mascherine di comunità riutilizzabili. L'igienizzazione accurata e frequente delle mani - è bene ricordarlo - è elemento essenziale della prevenzione del contagio, mentre l'uso dei guanti non previene in alcun modo il contagio ed è utile solo in particolari situazioni lavorative. Va promosso con decisione l'esame scientificamente fondato e assistito sulla presenza di virus o di materiale genetico di virus nelle acque reflue e del rapporto tra emergenza epidemiologica e inquinamento atmosferico, a partire dalle consapevolezze acquisite. La reazione a fatti illeciti e a possibili fenomeni illeciti dovrà avvenire sulla base del più ampio scambio di informazioni e di strumenti di coordinamento tra le autorità giudiziarie, polizia giudiziaria ed enti di controllo. La gestione dei rifiuti è sicuramente uno dei problemi più complessi del nostro tempo, in tema di ambiente e sicurezza. Secondo le varie disposizioni in materia, sia a livello mondiale che europeo e, infine, nazionale, si nota come sia necessario tutelare l'ecosistema e di conseguenza la salute dell'uomo, in vista di un'evoluzione culturale che porti alla progressiva diminuzione dei rifiuti. Con grande apprezzamento per i colleghi della Commissione - ricordo in particolare il presidente, onorevole Stefano Vignaroli e i relatori, il senatore Massimo Berutti e l'onorevole Giovanni Vianello posso affermare che la Commissione ha lavorato intensamente durante la fase emergenziale, audendo svariati soggetti, anche al fine di acquisire quante più informazioni utili possibili, volte alla produzione di una relazione che riuscisse ad essere esaustiva, sulla base delle evidenze scientifiche sin qui prodotte.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori, fino al 4 settembre. La seduta di domani avrà inizio alle ore 9, con la commemorazione del senatore Zavoli, recentemente scomparso. Seguirà la discussione del decreto-legge sulla parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario, già approvato dalla Camera dei deputati. Successivamente, il Ministro della salute renderà un'informativa sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19. I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti. Intorno al 18 agosto l'Assemblea sarà convocata per la comunicazione all'Assemblea del preannunciato decreto-legge recante misure economiche. I lavori delle Commissioni riprenderanno da lunedì 24 agosto, fatta salva l'autorizzazione a convocarsi anche in precedenza, in relazione a sopravvenute esigenze. L'Assemblea tornerà a riunirsi a partire da martedì 1° settembre, alle ore 16,30, con sedute fino a venerdì 4, se necessario, per la discussione del decreto-legge semplificazioni. Il calendario di tale settimana prevede, inoltre, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19 e il conseguente dibattito.

Invito i Capigruppo a verificare che gli interventi di fine seduta non siano ad esclusivo appannaggio dei soliti senatori, perché c'è una certa ricorrenza di taluni senatori e senatrici.

partito dalle università dell'isola e rivolto al titolare dell'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, Samonà. Si tratta di uno dei più antichi, cospicui e prestigiosi musei d'Europa, nato con il regio decreto del 17 giugno 1878, aperto nel 1886 e intitolato più tardi a Paolo Orsi, perché il celebre archeologo lo diresse dal 1895 al 1934. Dal 1977 è diventato regionale. Pensate che l'archivio storico e la biblioteca di questo museo avrebbero dignità di istituti autonomi, tanta è l'importanza delle attività e delle collaborazioni internazionali intrattenute con atenei e studiosi di grande prestigio, in centotrent'anni di vita. Paolo Orsi ha fatto ed è parte della storia dell'archeologia mondiale, punto di riferimento per la sua autorevolezza oltre che per la qualità dell'offerta, ma anche luogo di crescita per generazioni di ragazzi delle nostre scuole e straordinario campo di prova per moltissimi studenti universitari. Ciononostante, senza che sia riconosciuta la sua speciale dignità e il primato che gli spetterebbero anche per essere il museo più visitato dell'isola, oggi fa parte degli istituti del Parco archeologico di Siracusa, al quale l'assessore Samonà ha recentemente cambiato denominazione. Trattato nel contesto come uno fra i tanti, anche il museo Paolo Orsi rientra in quel terzo di musei italiani che dopo il *lockdown* non ha riaperto. Forse ricorderete che una funzionaria del museo è deceduta per Covid-19, ma voci di corridoio segnalano che la prolungata chiusura va imputata al fatto che l'edificio, situato nel parco Villa Landolina, aperto nel 1988 ma costruito nel ventennio precedente, soffrirebbe di importanti problemi strutturali non affrontati e di mancate manutenzioni. La miopia di un'amministrazione regionale da qualche tempo incapace di comprendere che investire denaro e risorse intellettuali nel museo Paolo Orsi significa assicurare all'isola intera progresso e ricchezza rischia di far sfumare le opportunità di crescita culturale ma anche economica offerte dal museo di Siracusa, peraltro da sempre all'avanguardia anche nell'impiego di nuove tecnologie in tema di visite guidate in presenza e da remoto. Nell'invitare tutti i colleghi e i cittadini italiani a firmare l'appello, anch'io mi rivolgo all'assessore Samonà per sollecitarlo a non legare il suo nome alla rovina del museo archeologico regionale Paolo Orsi, vanto della Sicilia, ma anche prestigioso tassello di storia della ricerca e della promozione del patrimonio culturale nazionale,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei attenzionare una storia appena iniziata ma che sono convinto proseguirà, vista la tenacia e la perseveranza degli attori protagonisti, in cui la solidarietà e la generosità umana danno il meglio di sé cercando di dare una risposta semplice, ma che viene dal profondo del cuore, ai bambini in difficoltà nel tentativo, riuscito, di regalare loro un sorriso e una gioia, considerate le loro complesse problematiche collegate allo spettro autistico. Questa patologia complessa, che questi piccoli pazienti condividono nella sua drammaticità con le loro famiglie, è di difficile approccio.

con scarso rispetto per l'Assemblea e soprattutto per lei, mi spiace ma proseguono. condividono con le loro famiglie è di difficile approccio terapeutico e di complicata risoluzione. La precocità e l'efficacia dell'intervento terapeutico in un percorso riabilitativo lungo e difficile riceve da questi momenti di intensa partecipazione e di uscita temporanea dal ritmo quotidiano una brusca accelerazione e una spinta estremamente positiva. Il gesto lodevole di Giuseppe, vigile del fuoco di Bari, che offre un giro in barca gratuito ai ragazzi autistici rappresenta un'iniziativa nobile, che dimostra da un lato il gran cuore e la generosità di chi l'ha promossa con semplicità e disponibilità, ma dall'altro anche la necessità e la forte richiesta d'aiuto, di una mano tesa e di una condivisione da parte dei ragazzi e delle loro famiglie così gravemente in difficoltà, ulteriormente accentuata dalla pandemia che abbiamo vissuto. Giuseppe ha messo a disposizione il suo gommone per regalare dei momenti di gioia a questi bambini e ragazzi autistici, con la speranza non celata che essi possano rappresentare per loro un piccolo aiuto capace di rompere il muro del silenzio e dell'isolamento che li avvolge, chiusi come sono nel loro mondo, ma con la voglia fortissima di aprirsi alla quotidianità.

da questo semplice gesto e aprirsi a iniziative realmente solidali e socialmente caratterizzanti! Occorre recuperare i valori profondi della solidarietà umana e sociale: facciamo sì...

Facciamo sì che l'iniziativa di Giuseppe non resti una goccia d'acqua nel deserto, ma apra a nuovi momenti e a provvedimenti capaci di portare a una... di porre sotto una luce nuova la problematica dell'autismo, ma anche le mille difficoltà che vivono le famiglie con figli autistici e i tanti risvolti, non solo clinici e riabilitativi, ma anche economici e sociali, che questa patologia comporta. signor Presidente, sottolineiamo sempre l'importanza di una precisa e ampia informazione, per allargare sempre di più la sensibilità e la condivisione di questa problematica da parte dei cittadini: l'autismo non è contagioso, l'ignoranza sì.

che può apparire marginale, ma non lo è e riguarda la questione della magistratura cosiddetta onoraria. È uscita di recente una sentenza di livello europeo che ha riconosciuto una dignità nella sostanza (e anche tante altre cose) ai magistrati onorari.

Ora, è bene che quest'Assemblea sappia che, in virtù di tale sentenza, in una materia delicatissima, com'è appunto la giustizia, lo Stato Italiano rischia - moltissimi contenziosi, soprattutto perché non è riconosciuta la dignità del lavoro, della funzione e dell'ufficio di questa magistratura. Nessuno naturalmente pensa che i magistrati onorari possano essere equiparati a quelli togati, non c'è una velleità di questo genere, vi è però un'esigenza,

Paese ed effettivamente il trascinarsi di questa questione è una specie di nuvola

quindi sia compito del Parlamento - e, in modo particolare, delle forze di maggioranza - non dimenticare questo tema,

che il *supermanager* commissario straordinario Arcuri ha fatto per la dotazione di banchi. La scadenza è stata prorogata dal 30 luglio al 5 agosto, quindi scade oggi. Nutro grandissime preoccupazioni, perché pare che il commissario straordinario non abbia ascoltato chi i banchi li produce. Nel bando sono previsti 3 milioni di banchi tradizionali, quindi quelli con i telai in acciaio, il piano in multistrato di betulla rivestito in laminato,

la quantità richiesta dei banchi tradizionali rappresenta la produzione normale di cinque anni, quindi si pretende che in tempi strettissimi delle aziende italiane facciano questa produzione, in un momento in cui, peraltro, c'è scarsità di acciaio,

un'impresa commerciale, che cercherà di raffazzonare, a destra e a manca, delle produzioni la cui qualità sarebbe tutta da verificare. L'anno scolastico inizierà scolastico inizierà senza che ci siano chissà quante centinaia di migliaia di insegnanti e con le scuole ancora non in sicurezza. Come sempre, questo Governo è arrivato tardi; il supercommissario, a braccetto con il Ministro, è arrivato tardi. A settembre le nostre scuole devono partire,

a dei lombardi, sempre con i piedi per terra, viene in mente: ma hanno fatto il conto che per consegnare, con il massimo ritardo l'8 settembre, tutte quelle produzioni

il mondo della scuola e le famiglie per un'ordinata ripresa dei lavori. Questo non è stato accettato e, quindi, mancheranno anche gli insegnanti e il balletto dei supplenti ricomincerà. Insomma, un fallimento completo. ahimè - temo di avere ragione. Il tempo per questo Governo e il supercommissario Arcuri è una variabile di poca importanza, mentre è di vitale importanza per noi, per le famiglie, per i Comuni e il Paese. *(Applausi)*. Consiglierei magari di prendere una piccola ripetizione da certi dirigenti dei Comuni che hanno già provveduto con tempestività a questi acquisti e alla sistemazione di tutto. Forse bisognerebbe ripartire dal basso per imparare qualcosa. *(Applausi)*.

grazie a tutti